l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti a tutti gli articoli

ancor prima dell'illustrazione degli emendamenti, mi limiterò a svolgere un intervento in termini assolutamente essenziali. evitato di esercitare la mia facoltà di replica, ma se da un lato è dovere del relatore, ove possibile, possibile, preservare la terzietà del proprio ruolo rispetto all'Assemblea è altrettanto vero che è diritto del relatore, quando è necessario, riportare il confronto e la discussione sui temi di merito, naturalmente rispettando ogni forma di dissenso rispetto al testo proposto, ma andando a contestare imprecisioni e inesattezze ovvero, quando ve ne siano, anche vere e proprie forme di ipocrisia. di ipocrisia. A tratti, nella discussione generale, alcuni richiami evocativi alle sette trombe dell'apocalisse o comunque a scenari allarmanti rispetto a questo provvedimento di legge esigono una replica. Non so se, nel caso specifico, l'ipocrisia sia realmente quella forma di omaggio e di rispetto che il vizio rende alla virtù; solo che mi è sembrato talvolta forzato andare a richiamare sforzi condivisi, pulsioni unanimi e poi argomentare, in un disegno di legge così delicato, di occasione perduta, quando per contro questo provvedimento di legge è un'occasione colta, valorizzata e portata fino in fondo. Questo provvedimento di legge, questo disegno articolato, ambizioso e prezioso va a colmare finalmente una straordinaria lacuna dell'ordinamento, va finalmente a regolamentare una materia delicatissima, va a raccogliere le puntuali indicazioni di tutti gli interlocutori istituzionali, va a valorizzare tutte le sollecitazioni qualificate che abbiamo raccolto in sede di Commissione giustizia al Senato. È un disegno di legge che vuole preservare la pienezza assoluta dei mezzi e degli strumenti di contrasto investigativo ad ogni forma di criminalità e di illegalità; ma vuole farlo conciliandola con la tutela estrema del diritto sacrosanto alla riservatezza di ogni cittadino, perché, Presidente, in uno Stato di diritto moderno l'unica sintesi possibile tra esigenze investigative ed esigenze di riservatezza

come si possa resistere rispetto alla riserva di giurisdizione, come si possa contestare la scelta di anticipare la giurisdizionalizzazione, di rafforzarla, di affidarla ad un giudice terzo che intervenga non soltanto nel momento dell'apprensione fisica dei dispositivi digitali, ma anche e soprattutto nella fase di accesso ai dati in esso contenuti, perché in una dinamica così delicata, così pericolosa, così pervasiva come l'accesso ai contenuti degli *smartphone*, dei dispositivi elettronici, in cui è racchiusa un'intera esistenza, vita, passioni, elementi personali, relazioni, che investe non soltanto l'ultimo detentore del dispositivo, ma tutta la rete di relazioni con la quale abbia, nel corso della vita, interloquito, un accesso privo di controlli e privo di regole assume una potenza devastante.

forse non l'unico possibile, ma nelle condizioni date - di questo sono convinto - il migliore possibile.

Signor Presidente, intendo chiarire le finalità dell'emendamento 1.200. In Commissione giustizia abbiamo tutti concordato sulla necessità di introdurre delle nuove regole per il sequestro dei cellulari, dei *tablet*, dei *computer* portatili per il motivo che questi apparecchi contengono una messaggistica - *chat*, SMS - che è parificata a corrispondenza e che quindi gode della tutela costituzionale di cui all'articolo 15. Per questo motivo, tutti abbiamo concordato sulla necessità che il pubblico ministero non può più autonomamente sequestrare questa apparecchiatura, ma deve richiedere l'autorizzazione del giudice. Senonché, quello che è accaduto è che la maggioranza, invece di tenersi dentro questo perimetro entro il quale vi era la concordia di tutti, ha ritenuto di dover debordare e quindi di estendere la nuova disciplina che si propone anche a documenti e dati che non hanno nulla a che spartire con il concetto di corrispondenza, perché in una memoria digitale, in uno *smartphone* possono trovarsi copie di fatture, di ricevute, di documentazioni bancarie e altri documenti che non sono assimilabili a corrispondenza e quindi non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione. Non solo, ma si è ritenuto di estendere questa nuova disciplina non solo al sequestro degli apparecchi di telefonia mobile, ma anche a memorie digitali, ad esempio a *pen drive* che non hanno nulla a che fare con il concetto di corrispondenza e che possono contenere, appunto, documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. A causa dell'estensione di questa nuova normativa anche ai dati che non hanno natura di corrispondenza e anche a memorie esterne e *pen drive*, si è creata una vera e propria schizofrenia nel nostro sistema processuale, perché si è creato un doppio regime normativo dei sequestri dipendente esclusivamente dalla natura del supporto del documento. anche quando sarà approvata questa nuova normativa resteranno in vigore le norme del codice di procedura penale che continuano ad autorizzare il pubblico ministero a sequestrare con decreto motivato tonnellate di documenti che non hanno natura di corrispondenza (contabilità aziendale, documentazione bancaria, ricevute e fatture). Questa norma Sennonché, se un pubblico ministero dovrà sequestrare anche una sola ricevuta in formato digitale, in *pendrive*, esclusivamente perché ha una natura digitale, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice, attivare un procedimento incidentale che prevede l'obbligo della notifica da un minimo di otto a un massimo di sedici persone (la persona indagata, quella offesa, quella a cui appartiene l'apparecchio, quella a cui dovrebbe essere restituita, i rispettivi avvocati), col pericolo che basta che soltanto una di queste notificazioni vada a vuoto perché occorra ricominciare da capo. Solo alla fine potrà effettuare il sequestro di questa sola ricevuta che si trova in un *pendrive*, col paradosso

non hanno natura di corrispondenza, dovranno attraversare questa procedura così complessa. Tra le ricadute vi è la diffusione del virus delle incompatibilità, perché avremo giudici che per sequestrare un *pendrive* in cui c'è una ricevuta diventeranno incompatibili a formare i collegi e quindi nei piccoli tribunali avremo la moltiplicazione delle incompatibilità e una paralisi. inoltre un inutile stress di uffici giudiziari, che già non hanno risorse, i quali dovranno distrarre fondi per fare decine e decine di notifiche per sequestrare documenti che non hanno nulla a che fare con la corrispondenza. Naturalmente questo servirà a tanti per traguardare l'agognato risultato della prescrizione e quindi dell'impunità. Con questo emendamento vogliamo quindi trovare una una razionalizzazione: spacchettiamo, distinguiamo il sequestro di tutti i documenti che hanno natura di corrispondenza da quelli che non hanno tale natura. Pertanto stabiliamo che, se devo sequestrare uno *smartphone,* chiedo una sola volta l'autorizzazione al gip per quanto riguarda i documenti quanto riguarda i documenti che non hanno natura di corrispondenza. Se dentro il cellulare, oltre alla corrispondenza, trovo ricevute, fatture e documenti che non hanno natura di corrispondenza, li sequestro senza bisogno di attivare quella procedura, così come li posso sequestrare in cartaceo. È una razionalità e serve a evitare una schizofrenia dell'ordinamento e uno spreco di risorse. È anche È anche una proposta di razionalizzazione che serve a raggiungere effettivamente il risultato di un ponderato equilibrio tra il diritto alla *privacy* e l'esigenza di efficienza delle indagini.

Signora Presidente, io illustro gli emendamenti anche per replicare alle considerazioni svolte dal relatore, ieri mi pareva di essere stato abbastanza chiaro nel mio intervento in discussione generale, quando ho spiegato noi siamo totalmente d'accordo sull'idea di introdurre una procedura giurisdizionalizzata per il sequestro degli *smartphone* nell'ambito delle indagini. Tanto è vero che siamo d'accordo che siamo stati forse quelli che più di altri, fin da subito, in esito all'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, hanno segnalato questa esigenza anche in ragione delle considerazioni fatte dal procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo. Questa posizione noi non la cambiamo. Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia necessario questo intervento. La nostra contestazione, che poi è stata riversata e tradotta in emendamenti puntuali, riguarda le modalità con le quali si è intervenuti, perché noi siamo convinti che si potesse fare - l'ho detto ieri e lo ribadisco adesso - un lavoro più accurato che non presentasse quei profili di criticità e di contraddizione che sono stati testé sottolineati dal collega Scarpinato, ma che anche noi non abbiamo mancato di far rilevare sia in discussione in Commissione, sia ieri in discussione generale. generale. Quelle contraddizioni e quelle criticità rischiano di mettere dei granelli di sabbia in una procedura, quella del sequestro degli *smartphone*, che merita di essere regolamentata e attribuita al controllo del giudice, ma che non deve essere resa difficile o farraginosa, perché se noi facciamo un procedimento che prevede una doppia richiesta, un doppio decreto e un doppio intervento del giudice, interventi sui quali si possono fare richieste di riesame, noi introduciamo una complicazione notevolissima nel procedimento, che rischia anche di innescare problemi non facilmente risolvibili nel caso in cui questo avvenga in uffici piccoli, dove i problemi di incompatibilità dei giudici che decidono sulle singole richieste di riesame rischiano di creare problemi insormontabili.

prendendo in considerazione per una volta in maniera più fattiva e costruttiva anche le ragioni e gli argomenti dell'opposizione non introducendo emendamenti all'ultimo minuto, come è stato in questo caso, che hanno completamente riscritto anche proposte di legge della maggioranza. Occorreva procedere in modo diverso per evitare questi rischi. I nostri emendamenti cercano di ricondurre alla linearità una proposta di legge, della quale noi condividiamo pienamente gli obiettivi e le finalità, ma che così redatta rischia di creare molti pasticci, oltre a restringere in maniera incongrua - e anche qui contraddittoria - il perimetro e l'area dei dei documenti sequestrabili attraverso il sequestro degli *smartphone*. Quindi, questa è la filosofia che ci ha ispirato. I nostri emendamenti sono finalizzati a questi obiettivi e a rendere più lineare ed eliminare le criticità del provvedimento, che sono figlie di questo modo di procedere, ma ci tenevo a ribadire che lo facciamo nello spirito costruttivo che ci ha animato in questo caso e che purtroppo la maggioranza non ha voluto cogliere. grazie.

L'articolo 2 prevede un emendamento che tiene conto della necessità, per evitare la paralisi degli uffici giudiziari, di aumentare il numero dei giudici, perché se abbiamo appena spiegato che quello che oggi si può fare con un decreto o con un'acquisizione del pubblico ministero, senza coinvolgere il giudice, cioè il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza, deve necessariamente passare attraverso una richiesta al giudice, perché oggi è tutto informatizzato e i documenti in cartaceo sono rari, questo significa che in ogni piccolo tribunale avremo la paralisi, perché quotidianamente i pubblici ministeri chiederanno ai giudici decreti di sequestro. Esauriremmo tutti i giudici possibili che non potranno più comporre collegi. Per questo motivo, tenuto conto che già c'è un'altra riforma che prevede il collegio per l'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare per la quale è stato proposto l'aumento dell'organico di 250 unità (assolutamente sottodimensionato rispetto alle esigenze), se si aggiunge questa ulteriore norma che prevede l'incompatibilità dei giudici, perché dovranno decidere quotidianamente su decine di sequestri di materiale che non è assimilabile a corrispondenza, dobbiamo necessariamente elevare almeno a 500 l'organico. Altrimenti questa sarà un'inefficienza programmata. Quando ai cittadini diciamo che i processi durano e che non possono concludersi entro breve termine, ciò non è frutto di un destino cinico e baro, ma di decisioni come queste, che mettono sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia *(Applausi)*, Qualcuno deve spiegare perché un pubblico ministero per sequestrare una ricevuta debba scomodare un giudice e paralizzare la giustizia. Aggiungiamo questo alla riforma della prescrizione e avremo il triangolo delle Bermude. Bermude. Attraverso queste tecniche defatiganti si disincentiva il ricorso ai riti alternativi e si arriva alla prescrizione dei reati in un Paese che in questo momento, a leggere la rassegna quotidiana del Ministero dell'interno, è una Caporetto della legalità, da Milano a Palermo. Invece di potenziare gli strumenti per la giustizia, cosa facciamo? Ci inventiamo procedure farraginose che non hanno alcun senso giuridico. Non c'è copertura costituzionale non viene in campo l'articolo 15 della Costituzione, perché dobbiamo scomodare un giudice per sequestrare una fattura. Qualcuno lo spieghi; non c'è alcuna spiegazione. Si chiama garantismo selettivo, che serve semplicemente a mettere sabbia negli ingranaggi della macchina della giustizia.

finestra"). Salutiamo e diamo il benvenuto agli studenti del Liceo di scienze umane «Giordano Bruno» di Roma e agli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Gian Domenico Romagnosi» di Erba, in Provincia di Como,

introduce una modalità di sequestro dei cellulari e dei *tablet* che è stata testata in alcune procure della Repubblica e che è idonea a garantire la tutela della *privacy* dell'indagato...

per garantire la tutela della *privacy* e l'efficacia delle indagini nel caso di sequestro di cellulari e di *tablet*. Sostanzialmente propone di estendere al sequestro di cellulari e di *tablet*, con i dovuti adattamenti, la stessa procedura che è prevista per le intercettazioni. Sottolineo che si tratta di un procedimento che è stato già applicato nella prassi

distinzione: il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione del giudice esclusivamente nei casi in cui debba sequestrare apparecchi elettronici che contengono al loro interno della corrispondenza, della messaggistica. caso, infatti, entra in campo l'articolo 15 della Costituzione che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Si prevede, invece, che il pubblico ministero, così come non deve richiedere al giudice l'autorizzazione per il sequestro di documenti che non hanno natura di corrispondenza - fatture, ricevute e documentazione bancaria - non debba richiedere al giudice l'autorizzazione anche quando questi documenti, invece che avere un supporto cartaceo, hanno un supporto informatico. Mi pare il minimo di razionalità. Non possiamo fare due regimi giuridici a seconda non della diversa natura del documento, ma del loro supporto. loro supporto. Si prevede che il pubblico ministero, effettuato il sequestro, immediatamente custodisca la copia informatica dell'apparecchio sequestrato nello stesso archivio digitale previsto per le intercettazioni. effettua immediatamente l'analisi del materiale rilevante per le indagini e procede alla distruzione di tutto quello che non è rilevante. Noi vorremmo sapere perché una procedura di questo genere debba essere bocciata e debba invece esserne prevista una complicatissima, che prevede la richiesta e l'autorizzazione del giudice anche per il sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza,

Chi ha proposto questo disegno di legge ha ascoltato le audizioni che si sono svolte in Commissione giustizia? Ha acquisito consapevolezza del qualsiasi cittadino che abbia un minimo di cultura informatica, un secondo dopo che gli hanno sequestrato un cellulare, va a casa, apre WhatsApp web sul computer e può cancellare immediatamente quello che c'è nel suo cellulare? Mettiamo quindici giorni di tempo a disposizione

WhatsApp mi pare follia, un regalo alla criminalità. Inoltre, questa proposta evita una seconda ricaduta negativa, e cioè quella di ingolfare gli uffici dei giudici con richieste di sequestro di memorie digitali che non contengono corrispondenza e che determinano l'incompatibilità successiva di quello stesso giudice che sequestra una memoria informatica a comporre i collegi giudicanti. Per questo insistiamo affinché venga votato il nostro emendamento.

questo intervento emendativo è un complemento del precedente: cerchiamo di limitare i danni. Invece di stabilire una procedura per cui entro cinque giorni il pubblico ministero deve attivare le notifiche a ben otto persone, come minimo,

e che il procedimento, invece di durare dieci giorni, abbia una durata di tre giorni. Ma cosa ci vuole a duplicare? È poi possibile che dobbiamo notificare all'indagato, alla persona offesa, al proprietario del telefonino, a chi ha diritto alla restituzione e - siamo a otto, se sono più imputati diventano sedici

Presidente, intervengo su questo emendamento, come potrei intervenire su altri, non per giustificare o per rendere ragione della nostra posizione, ma per esprimere, per oggi e per le prossime votazioni, il senso di disappunto che si prova quando un membro di questa Camera, peraltro ex pubblico ministero, si permette di parlare delle garanzie costituzionali per i cittadini con l'espressione che egli ha testé utilizzato nel generale disinteresse dell'Assemblea. Noi stiamo facendo queste norme per garantire ai cittadini il rispetto dei principi costituzionali della Parte I della Costituzione. *(Applausi)*. E Scarpinato usa il termine «malintenzionati», frutto di un giustizialismo di un giustizialismo che è ontologico, per cui il cittadino non è un cittadino che ha dei diritti costituzionalmente garantiti: per lui è un malintenzionato, uno di cui ancora non è stata provata la criminalità. Di questo si parla. Di fronte a questo atteggiamento culturale di Roberto Scarpinato, dei grillini e dei giustizialisti, mi stupisce il silenzio del PD, che non prende le distanze da un atteggiamento allucinante. Non sono malintenzionati: sono i cittadini, caro Scarpinato!

colleghi, nella mia esperienza di sequestri di cellulari e di materiale informatico ho purtroppo avuto a che fare con tanti malintenzionati che sono stati condannati con sentenza definitiva. Ho dovuto sperimentare che alcuni di questi malintenzionati sono stati capaci di alterare i dati sequestrati. Pertanto, non vi è alcuna volontà di offendere i cittadini, ma è un dato che traggo dalla mia esperienza.

che possa essere alterato da remoto, dobbiamo accelerare le operazioni di duplicazione. L'emendamento prevede pertanto che le operazioni di duplicazione debbano svolgersi nel più breve tempo possibile e non oltre le settantadue ore. Mi pare una garanzia per tutti

e ricordare a quest'Assemblea che i malintenzionati sono tali soltanto dopo il giudizio. Qui stiamo parlando di una fase molto preliminare nella quale, in questo momento, nel nostro Paese, vengono portati via degli strumenti che contengono tutta la nostra vita senza alcuna garanzia sia per chi sarà poi riconosciuto come malintenzionato, sia per chi sarà poi riconosciuto completamente innocente. Queste seconde persone come anche le prime, mi lasci dire - hanno tutte dei diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale e che in questo momento non sono efficaci. È veramente preoccupante una visione del diritto penale, per esempio, nella quale dice, soprattutto se ha un'esperienza come pubblico ministero e pubblica accusa, che sarebbe auspicabile sequestrare un telefono per poterci trovare all'interno un estratto conto. Mi viene da dire che, nell'esperienza di tutti noi, parte il fatto che, se la Polizia giudiziaria va in una banca e chiede l'estratto conto, le viene dato. Non c'è bisogno di andare a prendere un telefonino per fare una pesca a strascico. Si va nel luogo dove si può ottenere il mezzo di prova, con le maggiori con le maggiori garanzie possibili per l'imputato. Allora tu, Polizia giudiziaria, fai la fatica di andare a reperire l'estratto conto nella filiale di banca

vuole andare a pescare il malintenzionato - come dice il collega Scarpinato - ma nel rispetto delle garanzie costituzionali. Altrimenti entriamo in un'ottica del diritto penale nella quale, pur di condannare qualcuno, si fa strame delle garanzie costituzionali, nella visione secondo cui esistono non innocenti, ma soltanto colpevoli non ancora identificati; concezione del diritto penale che abbiamo conosciuto non solo, purtroppo, negli studi televisivi di questo Paese, ma soprattutto, dolorosamente, nelle aule di giustizia di questo nostro Paese.

Da vecchio psichiatra e antico politico vorrei capire, perché il termine mi spaventa molto per chi lo esprime, cosa significa in realtà "malintenzionato". È qualcuno che guarda l'anima di qualcuno in una profezia auto-avverante? O è il solito, riprovevole atteggiamento di chi vede il male potenziale in un altro, senza avere alcuna categoria scientifica né etica? A me questa cosa fa schifo e paura.

Il comma 10 del disegno di legge in esame prevede che, in alcuni casi di reati particolarmente gravi, si possa fare a meno della procedura di duplicazione, che abbiamo detto dura quindici giorni. In particolare, si fa riferimento ai procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis*, e 371-*bis*; si tratta di reati di mafia e di altri reati di questo genere. Noi proponiamo di inserire in questo elenco anche i reati del codice rosso e i reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

Prendiamo atto che non sono stati inseriti Senatore Licheri, confidi nella Presidenza. Anche lei, senatore Borghi.

Prego, il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Viviamo in un Paese in cui leggiamo ogni giorno, da Torino a Palermo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione *(Applausi)*, di comitati di affari, di cricche in combutta con i mafiosi,

Sì, però può darsi anche il contrario. alla collega Maiorino, per il suo tramite, che fintanto è vigente la Costituzione del 1948 tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva. *(Applausi)*. Non può essere, Tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e come tali vanno trattati, anche coloro... *(Commenti).*

Renzi, consentite alla Presidenza di tentare di regolare il dibattito. Intanto chiederei al vice ministro Sisto se può cortesemente riprendere

nella quale ci imbattiamo: far ricordare alla nostra opinione pubblica e anche agli illustri membri di questa Camera tutti gli imputati, anche quelli indagati per i crimini più odiosi, sono innocenti fino a sentenza definitiva. Non è che se io vengo indagato...

il fatto che sollevi ironie e battute il principio che tutti gli imputati sono innocenti fino a sentenza definitiva e che la gravità del reato del reato ascritto a una persona non è che lo renda un po' meno innocente, e quindi non è che la presunzione d'innocenza vale per il divieto di sosta e non vale per i reati di mafia. *(Applausi).* La presunzione di innocenza vale per tutti quindi, tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva. Ce ne dimentichiamo perché, per esempio, le nostre carceri sono imbottite, piene zeppe di gente che è in prigione prima della sentenza definitiva. *(Applausi)*.Siamo entrati in un'ottica della quale culturalmente e politicamente è soprattutto responsabile il MoVimento 5 Stelle - lo vediamo anche dal mercato del pesce indegno che è stato messo in scena questa mattina - per il quale per il quale la presunzione di innocenza in questo nostro Paese non vale più. *(Applausi. Commenti).* Mi faccia dire un'ultima cosa, signora Presidente: la presunzione di innocenza si applica anche a quelli che oggi stanno sulle prime pagine dei giornali.

La Presidenza insindacabilmente richiama i colleghi che stanno interrompendo inopinatamente il senatore Scalfarotto.

i malintenzionati, cioè i colpevoli di reati, vanno perseguiti, ma non a discapito delle loro garanzie costituzionali. Noi, pertanto, ci dobbiamo attrezzare questa la ragione per la quale, quando il senatore Scarpinato ha presentato emendamenti per l'assunzione di più magistrati, noi li abbiamo sempre votati. A nostro avviso dobbiamo mettere gli inquirenti in condizione di fare le loro indagini, ma non prendendo scorciatoie, non sacrificando i diritti dell'imputato. Va condannato il colpevole nel rispetto dei diritti costituzionali, perché questa è la Repubblica italiana. Quella che avete visto in scena in questo momento non è la Repubblica nata dalla Costituzione del 1948.

Supponiamo che un pubblico ministero ottenga dal giudice l'autorizzazione al sequestro di un cellulare di un'esponente della Guardia di finanza che abbia fatto un accesso abusivo per le segnalazioni di operazioni sospette e ottenga questo sequestro per reato di accesso abusivo. Poniamo che, effettuato il sequestro, esaminando le *chat*, accerti che quel poliziotto l'accesso abusivo l'ha fatto dietro la corresponsione di una somma di denaro da parte di terzo (reato di corruzione). Ebbene, il comma 14 di questo disegno di legge stabilisce che il pubblico ministero non potrà utilizzare quella *chat* per il reato di corruzione. Noi chiediamo, facendo ricorso alla sentenza Cavallo delle Sezioni unite della Cassazione, che almeno nei casi in cui vi sia una connessione tra reati,

perché quello che facciamo con questo ordine del giorno è semplicemente provare a portare lungo le linee logiche il disegno di legge e completarlo su alcune questioni che ci sembrano non non risolte. Quello che chiediamo, cioè, è che il contraddittorio e il potere decisionale del giudice delle indagini preliminari, quindi del giudice terzo, si applichino praticamente in ogni occasione, salvo casi assolutamente eccezionali. Proviamo a far diventare una regola quella per la quale, quando c'è un sequestro di un di un *device* tecnologico, di uno strumento tecnologico come un telefonino, il pubblico ministero e l'imputato - diciamo la parte contro la quale si procede - possano avere un contraddittorio davanti al giudice. Tra le altre cose, sempre nell'ordine del giorno, chiediamo di estendere le tutele a quella parte della messaggistica che c'è nel telefono, per esempio quella che intercorre tra il soggetto il soggetto proprietario dello strumento e il proprio difensore, che è un argomento del quale in Commissione ci siamo abbondantemente occupati dall'inizio della legislatura. Quindi, è un ordine del giorno e non un emendamento, perché non pretende di avere efficacia normativa immediata, ma chiede al Governo

Intanto la Presidenza è attenta, anche con la segnalazione dei senatori Segretari, che non ci siano voti che non corrispondano alla presenza.

Senatrice Fregolent, prima che lei intervenisse, questa Presidenza mi sembra che abbia già precisato con molta nettezza.

Dal giorno dopo l'entrata in vigore, il pubblico ministero che vorrà sequestrare documenti che non hanno natura di corrispondenza dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice, se questi hanno un supporto informatico. Questo determinerà l'incompatibilità di tali giudici a comporre successivamente i collegi giudicanti. Questo significa che nei piccoli tribunali, dove c'è un organico da venti a ventidue persone, si determina il pericolo di una paralisi. Se aggiungiamo che la riforma Nordio prevede un collegio per le ordinanze di custodia cautelare, ci rendiamo conto di trovarci dinanzi al pericolo di una paralisi degli uffici giudiziari, a meno che non si provveda, ora e non tra due anni, ad aumentare l'organico in modo congruo. Noi chiediamo che queste riforme, se devono camminare, camminino sulle gambe dei giudici che sono negli uffici e non determinino la paralisi degli uffici programmati. Se così fosse, noi ci troveremmo dinanzi a una inefficienza programmata, che lede il diritto dei cittadini ad un processo rapido ed efficiente.

Ogni qualvolta sono stati presentati emendamenti nei quali sono state chieste maggiori risorse, non solo per la magistratura, ma anche per il personale della della Polizia penitenziaria e per tutto il personale che lavora nelle carceri (psicologi, psichiatri o mediatori culturali), abbiamo sempre votato a favore e voteremo a favore. Non ci convince, Non ci convince, invece, l'idea che, dato che non ci sono sufficienti risorse, il prezzo delle carenze organizzative della giustizia si ribalti sulle garanzie costituzionali del cittadino. Quando sento dire che non si può fare l'udienza collegiale per la convalida del provvedimento di custodia cautelare perché non abbiamo abbastanza magistrati

Non è pensabile - dato che lo Stato non ce la fa a organizzarsi - limitare gli spazi di libertà dei cittadini. Allora, se ci vogliono più magistrati perché il processo sia equo, giusto e anche efficace (perché, lo voglio sottolineare, l'interesse alla repressione del crimine sta seduto su questi banchi come tra tutti gli altri banchi, anche quelli sotto i nostri), pensiamo soltanto che l'obiettivo a cui tendere, cioè quello di combattere la criminalità, non si possa risolvere, poiché non abbiamo gli strumenti, nel dire: cari cittadini, questo abbiamo e quindi voi, i vostri diritti costituzionali, li vedete ridotti. Questo non è pensabile. Pertanto, con la stessa energia, forza e determinazione con la quale abbiamo votato praticamente contro tutti gli emendamenti a questo disegno di legge, che ci pare un disegno di legge di civiltà,

aderiamo con convinzione e con convinzione voteremo a favore.

Colleghi, alle ore 14,45 il Presidente del Senato ricorderà le vittime dell'incidente di Suviana. Poiché è convocato il Consiglio di Presidenza, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,45.

riferiti a questo provvedimento, ci saranno fra poco le dichiarazioni di voto finali (sono iscritti i senatori Scalfarotto, Zanettin, Scarpinato, Erika Stefani, Verini

Cari senatori e care senatrici, come sapete, purtroppo ieri una violenta esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese, ha provocato

minuti fa, della situazione. Lo scenario, come mi è stato riferito, è tuttora molto critico e anche pericoloso. Mentre vi parlo, i soccorritori - a cui rivolgo il mio e il vostro sincero sincero ringraziamento - sono ancora impegnati nelle operazioni, in condizioni difficilissime. Quella di Suviana è l'ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro: ancora una volta, vite spezzate laddove ci si reca per lavorare. Questo è un dramma enorme, che continuiamo a vivere quasi ogni giorno. Quella di Suviana

di intervento immediato, capire fino in fondo cos'è successo. Nonostante negli anni siano stati diversi gli aggiornamenti al sistema normativo, tuttavia ci troviamo ancora oggi a commemorare dei morti. Avere più sicurezza è un impegno difficile, lo sappiamo bene; ma non è, non può essere e non deve essere un impegno impossibile. Occorre però la volontà di tutti, nessuno escluso, dalle istituzioni, centrali e locali, e dalle imprese ai lavoratori stessi, passando infine per le figure preposte al controllo della sicurezza: ognuno deve fare la propria parte. Desidero, care senatrici e cari senatori, formulare in quest'Aula il cordoglio personale e quello del Senato alle famiglie delle vittime e gli auguri di pronta guarigione agli operai rimasti feriti. La nostra sincera vicinanza va inoltre alle famiglie dei dispersi e la loro speranza è è anche la nostra speranza e il dolore di tutte le famiglie di chi è rimasto coinvolto è anche il nostro dolore. Vi chiedo di osservare qualche attimo di silenzio.

Voglio ricordare anche i due Carabinieri morti nell'incidente stradale nel Salernitano, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferrara. All'Arma dei Carabinieri e ai familiari dei due militi vanno la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.

Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Italia Viva - Il Centro - RenewEurope per annunciare - lo dico sin dall'inizio - il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Il nostro convinto a favore di una norma che penso abbiamo atteso anche per troppo tempo. La nostra legislazione fa fatica a star dietro agli sviluppi tecnologici e ai cambiamenti rapidissimi del nostro modo di vivere una questione che sicuramente avevamo aperta davanti agli occhi è quella del nostro rapporto con questi strumenti tecnologici che ormai, come tanti colleghi anche durante la discussione generale hanno detto, sono diventati veramente parte integrante delle nostre vite, quasi un prolungamento delle nostre mani, dei nostri occhi e delle nostre teste, soprattutto i telefoni cellulari. Questi strumenti contengono al loro interno sostanzialmente tutta la nostra vita, perché dentro un telefono cellulare ci sono ovviamente tutti gli indirizzi delle persone che conosciamo e le nostre fotografie dei nostri momenti privati; attraverso l'utilizzo del telefono cellulare possiamo sapere

i dati della salute di una persona; i nostri conti correnti ormai sono praticamente dentro il nostro telefono cellulare, tramite il quale possiamo sapere quanti soldi ci sono nel conto corrente, quali sono gli investimenti fatti da una persona o i pagamenti che ha eseguito. Oppure, non avete mai pensato ai nostri acquisti *online*? Il profilo come consumatore di ognuno di noi è determinato dal fatto che si compra sempre più *online* e sul vostro *account* di Amazon si saprà se vi piace comprarvi un paio di scarpe anziché un altro, che libri leggete o che musica ascoltate. È chiaro quindi che intorno a quegli strumenti è necessario stabilire una rete di protezione, che è quella che i nostri costituenti e il legislatore fino ad oggi consideravano propria della

Da quanto tempo - mi viene da chiedervi, colleghi e colleghe - non comprate un francobollo e non spedite una lettera cartacea? Oppure, mi viene da chiedervi quanto oggi telefonate a voce e quanto scrivete su WhatsApp. Ci pensavo ieri, ascoltando il collega Bazoli, quando diceva state allargate alla messaggistica le stesse norme delle intercettazioni. Penso che sia giusto. Non so cosa capiti nella vostra esperienza, ma di telefonate a voce

Erano finanziatori di una fondazione politica, il cui nome è Open, e tutti contributori tramite fondi che erano versati assolutamente in modo trasparente attraverso bonifici bancari, bonifici bancari, che - mi viene da dire - erano facilissimi da reperire, perché bastava andare in banca, chiedere l'estratto conto della fondazione Open e sarebbero risultati tutti. Invece si prendono Invece si prendono questi strumenti, che contengono tutte le cose di cui vi ho parlato sin qui, e vengono portati via ai legittimi titolari, le cui vite, ben al di là di quel singolo finanziamento fatto alla Open, sono state nelle mani degli inquirenti e purtroppo, come accade spesso nel nostro Paese, sono finite sui giornali: tutto. Mi si viene a dire che dobbiamo essere pronti a

che è fatta da magistrati, i più alti magistrati del Paese, che hanno detto chiaramente alla procura di Firenze che quei sequestri erano illegittimi. Vi leggo parole scritte dalla Suprema corte di cassazione: si trattava di una ricerca di dati esplorativa e sproporzionata, di un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali; si trattava - dice ancora la Cassazione - di un sequestro strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva. Cinque volte la Corte di cassazione afferma che quel sequestro era sbagliato, fatto male, ingiusto e ingiustificato, parlamentari del Senato ha dovuto riconoscere, praticamente quasi all'unanimità (diciamo a larghissima maggioranza), che quelle cinque sentenze della Corte di cassazione costituivano *fumus persecutionis* nei confronti di un parlamentare. Mi viene da dire: se quella persona non fosse stata un parlamentare? Se non avesse avuto gli strumenti che ha un parlamentare, che tipo di tutela avrebbe avuto in una situazione del genere? genere? Io credo che queste tutele vadano riconosciute a tutti. Bisogna che torniamo - e orgogliosamente - nell'alveo della presunzione di innocenza. Dobbiamo recuperare la cultura delle garanzie del processo

il potere coercitivo dello Stato, che si ferma davanti alle garanzie riconosciute all'imputato. Le nostre democrazie nascono da lì.

quello che sto dicendo in una sentenza che, appunto, dice che quella messaggistica equivale a corrispondenza e non a semplice documentazione. Questo disegno di legge in fondo fa questo e lo fa anche in modo ragionevole, perché, per esempio, stabilisce che, in caso di urgenza, sia ancora il pubblico ministero a occuparsi di queste incombenze, anche se ovviamente con le garanzie dell'intervento del gip. Noi ci siamo permessi, con convinzione, di presentare un ordine del giorno che malauguratamente la maggioranza e in questo fa sempre capolino quel dualismo tra garantismo e "manettarismo" che contraddistingue questo Governo - non ha accolto. Avremmo voluto un maggiore coraggio per definire in modo completo il ruolo del giudice delle indagini preliminari che, in quanto terzo e imparziale, nel quadro di un processo accusatorio, deve mettere le due parti in una situazione di piena parità. Il Governo non lo ha fatto, ma comunque pensiamo che questo disegno di legge rappresenti un grande passo avanti. Si era capito che serviva, anche all'esito dell'importante indagine conoscitiva che abbiamo fatto in Commissione giustizia, e devo dire che sulla necessità di questo disegno di legge

voluta da questa maggioranza di centrodestra, in particolare da Forza Italia, come elemento qualificante della nostra azione politica. Si deve ricordare che nel primo anno di questa legislatura la Commissione giustizia del Senato, su impulso della presidente Bongiorno, ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, al fine di evidenziare le criticità e i possibili interventi normativi per meglio bilanciare, in chiave garantista, i rapporti tra difesa e pubblica accusa, che sono stati alterati negli ultime legislature a seguito di legislazioni manettare e giustizialiste. Da tale poderoso lavoro è emersa, tra le altre cose, la necessità di questo disegno di legge e di una disciplina del sequestro dello *smartphone*, che, a fronte di una sempre più sofisticata digitalizzazione della società, contemperasse le obiettive esigenze delle indagini, per accertare e punire chi commette reati, assicurandolo alla giustizia, con la tutela della *privacy* dei cittadini, che - ricordiamolo - è un diritto primario di rango costituzionale, protetto dall'articolo 15 della Costituzione. Il tumultuoso progresso tecnologico ha trasformato infatti il telefono cellulare, lo *smartphone* che tutti adoperiamo e portiamo con noi, nella scatola nera della vita di ciascuno. Nello *smartphone* finiscono registrati non solo i contatti telefonici, le *chat* delle applicazioni di messaggistica e le *email*, ma anche le foto, i video della vita privata, i dati sanitari, fiscali, bancari, talvolta anche registrazioni della sfera intima. Nello *smartphone* finiscono però anche i dati di terzi, perché ormai questi strumenti sono diventati anche sostituti delle relazioni interpersonali, che sempre più si svolgono attraverso scambio di messaggi scritti o vocali. Acquisire in modo massivo i contenuti di un telefonino significa quindi violare e travolgere la *privacy* non solo dell'indagato, ma anche di soggetti terzi del tutto estranei alle indagini. Ad oggi, colleghi, nessun atto investigativo è invasivo della *privacy* di un indagato e di coloro che con lui abitualmente interagiscono quanto il sequestro dello *smartphone*, che ha la capacità di mettere letteralmente a nudo l'universo mondo dei soggetti coinvolti. Le tradizionali intercettazioni telefoniche o ambientali non hanno mai avuto nel nostro ordinamento una pervasività nemmeno paragonabile. paragonabile. A fronte della prodigiosa evoluzione tecnologica, le norme codicistiche del sequestro penale appaiono obsolete ed inadeguate e necessitano di una revisione.

Il sequestro di *smartphone*, in relazione ai dati altamente sensibili in esso contenuti, necessita pertanto di disciplina *ad hoc* e dovrà essere quindi circondato da garanzie paragonabili piuttosto a quelle proprie delle intercettazioni rispetto a quelle tradizionali del sequestro probatorio. La selezione dei loro contenuti dovrà poi essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni, e cosa invece non è penalmente rilevante, deve rimanere segreto, non transitare nel fascicolo del dibattimento e tantomeno finire sulle pagine dei giornali. Ciò è esattamente quanto è previsto da questo nostro disegno di legge, che propone di introdurre l'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale, prevedendo una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, prevedendo, riguardo riguardo alla procedura, che l'autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione all'oggetto delle indagini, con criteri di proporzionalità e adeguatezza. Originariamente, il disegno di legge a mia prima firma prevedeva che a disporre se questo fosse il pubblico ministero. Molto opportunamente - io credo - il relatore, senatore Rastrelli, che ringrazio per l'accurato e approfondito lavoro svolto in Commissione, ha delineato con una riformulazione una procedura diversa e ancora più garantista di quella ipotizzata nella prima stesura.

nella quale, a maggior garanzia dell'indagato e dei terzi coinvolti nei contatti, è chiamato ad esprimersi un giudice e non solo il rappresentante della pubblica accusa. Anche il giudizio sulla penale rilevanza dei dati da acquisire al fascicolo è di competenza del gip. Sulla giurisdizionalizzazione del procedimento mi pare siano ora d'accordo - almeno così ho colto dagli interventi sia in discussione generale che questa mattina nell'illustrazione degli emendamenti - anche le opposizioni. Va ribadito che ciò che è penalmente rilevante deve rimanere nell'archivio segreto, non deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento né tantomeno divulgato a terzi o, peggio, ai *media*. signor Presidente, perché sottolineo in modo così netto e preciso la necessità di mantenere segreti i dati acquisiti con il sequestro dello *smartphone*. Poco fa il senatore Scalfarotto nel suo intervento ha parlato di un caso di vita vera. Anch'io, suo tramite, signor Presidente, al senatore Scalfarotto parlerò di un caso di vita vera e concreta. Il sottoscritto è stato in passato indirettamente interessato dal sequestro di un telefonino di un soggetto terzo.

La mia *chat* con Luca Palamara non aveva né ha mai avuto rilevanza penale né tantomeno disciplinare, né tantomeno per così dire "gossippara", al punto che nessun *media* l'ha mai né commentata né rilanciata. Aveva contenuti esclusivamente istituzionali e di circostanza. Ciò nonostante, questa *chat* ancora oggi è pubblica, in quanto prima oggetto di un sequestro, poi acquisita al fascicolo di indagine, transitata quindi sulle pagine dei giornali e infine *online*. Non ho mai fatto una questione politica di ciò, anche se riguardava un periodo nel quale ero pure parlamentare e quindi protetto dalle speciali guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione, ma credo che ciò sia stato comunque un fatto ingiusto ed esagerato. In quella vicenda, molto peggio è andata a tanti magistrati interlocutori di Palamara. Le loro *chat*, dichiarate penalmente irrilevanti, dichiarate disciplinarmente irrilevanti, giudicate irrilevanti anche sotto il profilo della incompatibilità in prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, divenute pubbliche, però, sono state utilizzate impropriamente per penalizzare prospettive di carriera, mortificare professionalità, esporre alla gogna mediatica. Talune contenevano espressioni gergali, confidenze improprie, talvolta addirittura epiteti scurrili, poco confacenti alla funzione, ma sono convinto dovessero comunque rimanere segrete, coperte dalla tutela dell'articolo 15 della Costituzione, e che sia stato un abuso divulgarle. Con questo intervento normativo si potrà dunque porre finalmente un freno a scempi di tale natura. Ho ascoltato con attenzione le critiche che sono state portate a questo provvedimento nel corso della discussione generale e nel dibattito di questa mattina. Non mi convince, senatore Scarpinato, chi critica le maggiori garanzie per il cittadino indagato previste da questo disegno di legge. Io replico che le garanzie non sono mai troppe, se sottese alla tutela di principi di rango costituzionale, come il diritto alla *privacy* e la presunzione di non colpevolezza. Non mi pare pertinente neanche l'esempio citato, sempre dal senatore Scarpinato, ma anche dal senatore Bazoli, con riferimento all'ipotesi di reato contestata al finanziere responsabile di un presunto dossieraggio ai danni di politici piuttosto che di uomini e donne dello spettacolo. Nel caso specifico, per il reato di cui all'articolo 615-*ter* del codice penale, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dell'agente e dall'accesso ad una banca dati di pubblico interesse, la pena prevista varia da un minimo di anni tre al massimo di anni otto e giustifica quindi, anche *de iure condendo*, sia le intercettazioni telefoniche che il sequestro di *chat* e *mail*. L'approvazione di questo disegno di legge, come sottolineato da molta dottrina, è urgente e, per certi versi, addirittura tardiva, perché di fatto va a recepire un'evoluzione giurisprudenziale già matura, che si ispira in particolare alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e a diverse sentenze della Corte di cassazione. In conclusione dell'intervento voglio ringraziare il vice ministro Sisto per il proficuo lavoro svolto in Commissione, sempre a supporto della nostra iniziativa legislativa, che si colloca nell'alveo della poderosa riforma della giustizia di stampo garantista, cui Forza Italia lavora e i cui contorni si stagliano sempre più nitidamente in questi mesi. Come ieri è stato ricordato in discussione generale in Commissione giustizia, stiamo per approvare un nuovo testo della disciplina della proroga delle intercettazioni, che pure è stato ispirato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia. Nel disegno di legge Nordio, già votato in questo ramo del Parlamento e di prossima approvazione alla Camera, è stato trasposto il divieto assoluto di intercettazioni delle conversazioni tra avvocato e cliente, che pure era stato ispirato dalla stessa indagine conoscitiva. In Commissione giustizia voteremo a breve anche la riforma della prescrizione, che tornerà ad essere un istituto di diritto sostanziale. Insomma, rimane solo la separazione delle carriere, alla quale Forza Italia tiene molto, ma che il ministro Nordio ha annunciato passerà a breve al vaglio del Consiglio dei ministri. Un ringraziamento non formale lo voglio rivolgere anche alla presidente Bongiorno Bongiorno per l'autorevolezza con cui guida la nostra Commissione, a tutto il personale della Commissione giustizia, ai funzionari di Commissione e dell'Ufficio studi, che ci supportano sempre con grande professionalità e competenza nella nostra opera di legislatori.

Signor Presidente, nell'esordio di questa dichiarazione di voto, io tengo a sottolineare che il MoVimento 5 Stelle è stato il primo partito, in ordine temporale, che ha depositato, il 9 maggio 2023, un disegno di legge, a mia firma, per introdurre, nel codice di procedura penale, una nuova disciplina del sequestro dei dispositivi di comunicazione mobile, cellulari, *tablet* e *personal computer*. Depositammo quel disegno di legge ritenendo indispensabile che il legislatore intervenisse con urgenza su questa materia, per due ordini di motivi. In primo luogo perché questi apparecchi contengono messaggistica di varia tipologia - *chat*, *mail* sms - che, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, va qualificata come corrispondenza la cui libertà e segretezza è presidiata all'articolo 15 della Costituzione. Dunque il sequestro deve essere autorizzato dal giudice e non può essere disposto autonomamente dal pubblico ministero. In secondo luogo perché il regime normativo attuale autorizza il sequestro indiscriminato di tutto il contenuto degli apparecchi sequestrati e non imponendo la successiva secretazione della parte di questo contenuto che non è rilevante per le indagini, determina una violazione del diritto alla riservatezza che non è necessitata da esigenze investigative, ma è causato soltanto da un *deficit* normativo. Per ovviare a questi gravi limiti, il nostro disegno di legge proponeva una nuova disciplina legislativa che prevedeva una sequenza procedimentale semplice, rapida, lineare, già felicemente sperimentata in alcune procure della Repubblica e idonea a bilanciare la tutela della riservatezza con l'efficacia delle indagini. In sostanza, si proponeva di estendere al sequestro dei cellulari e dei *tablet* la stessa disciplina delle intercettazioni, con opportuni adattamenti. In sintesi, si prevedeva che il pubblico ministero non potesse più procedere autonomamente a questi sequestri, ma dovesse richiedere l'autorizzazione del giudice. Effettuato il sequestro, il pubblico ministero doveva, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore, realizzare una copia del contenuto dello strumento sequestrato con una procedura idonea ad assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Questa copia doveva essere immediatamente conservata nell'archivio digitale delle intercettazioni, che come sapete è coperto dal segreto d'ufficio; il pubblico ministero doveva selezionare rapidamente gli elementi utili per le indagini e distruggere della copia che non era rilevante per le indagini. Ingenuamente, ci attendevamo che su una simile proposta potessero convergere, con eventuali integrazioni o modifiche, tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza già nel maggio dell'anno scorso, facendosi carico comune della necessità condivisa di dare risposta rapida alle esigenze dell'amministrazione della giustizia dei cittadini. Ma si trattava, per l'appunto, di un'ingenuità e di un'illusione, perché, cammin facendo, nel corso di questa legislatura, abbiamo dovuto prendere atto che questa maggioranza, nel realizzare le riforme sulla giustizia, antepone sistematicamente agli interessi generali della collettività e della giustizia, l'interesse particolare di limitare, ostacolare e imbrigliare in tutti i modi possibili i poteri di indagine della magistratura nei confronti dei reati dei colletti bianchi, strumentalizzando a questo fine tutte le occasioni che si presentano e celando questo obiettivo dietro complessi tecnicismi che non sono comprensibili al cittadino medio e dietro la maschera di un garantismo di mera facciata. Per ragioni di tempo, mi limiterò a due esemplificazioni di come questa tecnica legislativa di strumentalizzazione occulta delle riforme sia stata realizzata anche nel disegno di legge in esame. Il primo esempio è legato alla più recente attualità ed è immediatamente comprensibile anche dai senatori che non hanno competenze giuridiche: poniamo che una procura della Repubblica individui alcuni esponenti delle Forze di polizia che hanno effettuato migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti personaggi politici sensibili e importanti esponenti del mondo imprenditoriale e che il pubblico ministero chieda e ottenga dal giudice il sequestro dei cellulari e dei *tablet* degli indagati per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e per il reato di abuso d'ufficio. Poniamo che a seguito dell'esame del materiale sequestrato, il pubblico ministero individui *chat* e *mail* che attestano che quegli accessi abusivi sono stati effettuati su richiesta di terzi dietro corresponsione di somme di denaro, prove inequivocabili del reato di corruzione previsto dall'articolo 319. Oggi, con l'attuale normativa, il pubblico ministero può utilizzare queste *chat* per procedere anche per reato di corruzione. Ebbene, dal giorno successivo all'approvazione di questo disegno di legge il pubblico ministero sarà privato della possibilità di utilizzare le *chat* che provano la corruzione. Il comma 14 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede infatti che i materiali sequestrati non possano essere utilizzati per reati diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati i sequestri, tranne che per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, tra i quali, come è noto, non rientrano i reati di corruzione e altri reati dei colletti bianchi. E questo neanche nei casi in cui un reato, la corruzione, sia stato commesso per eseguire un altro reato, l'accesso abusivo ai sistemi informatici. Un esempio paradigmatico di come questa maggioranza approfitti di ogni occasione per mettere sabbia negli ingranaggi del contrasto alla corruzione. Un esempio paradigmatico di garantismo classista, utilizzato alla bisogna come alibi per garantire l'impunità di classe dei colletti bianchi dalla stessa maggioranza, pronta a tramutarsi in feroce giustizialista per i reati della gente comune e degli emarginati, prevedendo l'utilizzo a tutto spiano di intercettazioni e di *trojan* per reati come i *rave party* e, da ultimo, persino per il reato di induzione all'accattonaggio, come proposto dall'articolo 13 del pacchetto di sicurezza presentato alla Camera il 12 gennaio 2024 dai ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio. L'induzione all'accattonaggio sì, la corruzione no: se questa non è giustizia di classe, cos'è la giustizia di classe? Non lo so. Per ragioni di tempo mi devo limitare solo a un altro esempio della finalizzazione occulta di questo disegno di legge, quella di imbrigliare i poteri di indagine del pubblico ministero senza valide ragioni. Il codice di procedura penale vigente attribuisce al pubblico ministero il potere di sequestrare, con decreto motivato, i documenti e i dati che non sono in alcun modo assimilabili al concetto di corrispondenza, per esempio fatture, documentazione bancaria e aziendale, fotografie, eccetera. Questo disegno di legge priva il pubblico ministero di questo potere quando questi documenti sono su supporto informatico, ad esempio quando sono contenuti in una *pen drive*. In questi casi, anche se si tratta di documenti che non sono coperti dall'articolo 15 della Costituzione, il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione al giudice, deve dare vita a un procedimento incidentale per la duplicazione del supporto, con la notifica ad almeno otto soggetti, che possono diventare e infine, nella terza fase, può fare il sequestro. Un vero e proprio sfiancamento delle indagini, che determina un enorme spreco di risorse e di tempi. Si consideri che è sufficiente che una sola di queste numerose notifiche vada a vuoto, perché si determini la necessità di ricominciare da capo. Si consideri l'effetto perverso della diffusione a catena del virus delle incompatibilità, perché il giudice che ha autorizzato il sequestro di una *pen drive* diventa incompatibile a formare i collegi giudicanti. Si consideri l'assurdo giuridico per cui questa complessa procedura è prevista solo se i documenti sono su supporto informatico, mentre, se sono su supporto cartaceo, il pubblico ministero non ha bisogno di attivarla e può sequestrare direttamente Mi avvio alla conclusione. Un altro piccolo capolavoro di ingegneria giuridica, non giustificato da alcuna valida ragione istituzionale, ma idoneo a contribuire ad ingolfare ulteriormente, con una miriade di defatiganti adempimenti, uffici giudiziari che sono già allo stremo per carenza di mezzi e di risorse, allungando a dismisura i tempi del processo e offrendo così a tanti l'ancora di salvataggio di traguardare i tempi di salvifiche prescrizioni. In questo Parlamento - e qui concludo - sembra di vivere in un'altra Italia. Mentre il Paese reale è dissanguato, da Nord a Sud, da un esercito di cricche, di comitati d'affari in combutta con clan mafiosi, nelle Aule parlamentari, dall'inizio di questa legislatura, la principale preoccupazione della maggioranza di Governo non è quella di contrastare la corruzione e la mafia dei colletti bianchi, ma, al contrario, quella di contrastare la magistratura, gli organismi di controllo e il giornalismo investigativo indipendente. Non possiamo che prendere atto che in Parlamento convivono e si confrontano le rappresentanze politiche di due Italie diverse: quella dei potenti intoccabili e quella dei cittadini che credono ancora nella giustizia e nella legalità. E siccome noi rappresentiamo questi ultimi, non voteremo questo disegno di legge.

di riprendere dei concetti di garanzia e di tutela che magari nel tempo si sono venuti un po' ad incrinare. Si vive un periodo abbastanza particolare, nel quale pare che vi sia una contrapposizione fra politica e magistratura, contrapposizione alimentata, in realtà, da alcuni Gruppi politici che probabilmente su questo intendono fare campagna elettorale e recupero di consensi, quando invece noi vogliamo semplicemente ristabilire i poteri e la stessa separazione dei poteri.

interessi che paiono anche contrapposti, ma che vanno a incidere su temi e diritti meritevoli di tutele anche costituzionali. Ci siamo accorti un po' tutti - diremo in particolare dove - di questa lacuna che si era trovata all'interno dell'ordinamento. Infatti, se per un verso sul tema delle intercettazioni si è legiferato, si è intervenuti, si è cercato di

perché i tempi sono cambiati: ormai la corrispondenza non è più la lettera cartacea firmata e mandata per posta;

che si è conclusa con un documento condiviso a larga maggioranza, ma probabilmente alcuni temi sono stati più condivisi di quanto non abbia dimostrato il voto finale, perché soprattutto sul tema del sequestro di documenti informatici abbiamo avuto una larga condivisione anche da parte della stessa Commissione. Ricordo qual è il tema che abbiamo sottolineato. Intanto, è stato sollevato un problema sulla garanzia dei contenuti del sequestro di dispositivi e dei contenuti che non sono particolare oggetto delle indagini. Ciò perché se, per un verso, le captazioni nel sistema delle intercettazioni hanno delle garanzie procedimentali e presentano anche una forte tutela della riservatezza, in quanto è previsto l'archivio riservato,

Ci sono, infatti, degli interessi contrapposti: uno è quello che va dall'accertamento dei fatti all'acquisizione della prova, l'altro è il diritto non solo alla dignità e alla reputazione della persona, ma anche alla libertà stessa dell'individuo.

diritti fondamentali ed è per questo che si chiede l'intervento del gip. Ricordiamo che questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare e anche questo è un aspetto importante che sottolinea ancora l'importanza del Parlamento, che quindi si tira fuori da quel ruolo, di cui a volte è stato

parlando in particolare del caso che riguardava il senatore Renzi e anche l'applicazione delle guarentigie parlamentari, ma che pone anche un altro tema. Per esempio, se io

L'attività investigativa non deve seguire i principi del *whatever it takes*, che ci piacque in altri settori, ma che nel caso di una indagine investigativa non obbedisce ai princìpi di una civiltà Non siamo qui per difendere le posizioni di una singola persona o la storia personale di chi ha subìto la pubblicazione di alcune intercettazioni, di chi ha subìto dei processi che alla fine si sono chiusi con delle assoluzioni, ma siamo qui

vorrei segnalare un dato politico che - secondo noi - attiene al rapporto che questo Governo, questa maggioranza, hanno con il sistema della giustizia e che - non giriamoci attorno - si è palesato con evidenza in molti dei provvedimenti che abbiamo affrontato negli scorsi mesi, dalla prescrizione all'abuso d'ufficio, dai test psicoattitudinali per i magistrati agli attacchi - secondo noi - all'autonomia della magistratura. L'elenco potrebbe essere più lungo, perché un assillo di questo Governo sembra essere quello di indebolire l'azione della magistratura, la sua indipendenza, colpendo il principio civile e costituzionale della separazione dei poteri, o quantomeno quello di rendere più complicato, più difficile il lavoro della magistratura, soprattutto nel contrasto e nel perseguimento di alcuni tipi di reati. Questo provvedimento ne è un esempio. Lo ha detto bene ieri il senatore Bazoli: questa avrebbe potuto essere un'occasione per un lavoro comune, giungere a un esito condiviso con convergenze larghe. C'era il disegno di legge a doppia firma Zanettin-Bongiorno e c'era l'altro disegno di legge del senatore Scarpinato: erano basi importanti, nella sostanza condivisibili. Invece non avete voluto, non siete stati in grado di cogliere questa opportunità. Respingendo tutte le osservazioni e gli emendamenti che anche l'opposizione nel suo insieme ha prodotto, siete stati in grado di compiere un pasticcio, anche in un provvedimento come questo che era partito su binari accettabili. Del resto, erano state le parole del ministro Nordio, qualche mese fa, a essere chiare: collegandosi a questa norma, si spinse a dire come sia inaudito che uno *smartphone* possa essere sequestrato con la sola firma di un pubblico ministero, vista la concentrazione di notizie che possono essere in esso contenute. Insomma, per il ministro Nordio, con un richiamo che noi consideriamo in questo caso improprio alla Costituzione, il sequestro fatto dal singolo magistrato confliggerebbe con qualsiasi regola. Sappiamo tutti - e voi lo sapete certamente meglio di me e lo dico davvero - quanto l'oggetto *smartphone* sia un simbolo di questo tempo. In questi apparecchi - è vero, lo sappiamo - c'è la vita, quasi tutta la vita di tante persone - ciò la dice lunga - e in particolare di tanti giovani. Ci sono sogni, speranze, segreti d'amore ed affetti. Spesso è un antidoto - spesso un falso antidoto, ma comunque un antidoto - a solitudini e crisi esistenziali. E le cose intime, personali vanno tutelate. Non si tratta quindi, ovviamente, di mettere in discussione la riservatezza dei dati a disposizione del magistrato, la tutela della *privacy* per i diretti interessati, oltre la fattispecie degli eventuali reati su cui si sta indagando. La tutela della *privacy* e la riservatezza vanno rispettati, però sempre e non a corrente alternata. Lo dico senza *vis* polemica particolare: i dati riservati da proteggere possono e debbono essere certi dati contenuti in questi strumenti, ma potevano essere anche quelli dei rappresentanti della Polizia penitenziaria di Sassari, che un sottosegretario come Delmastro ha invece diffuso. Erano dati riservati anche quelli. I dati riservati vanno tutelati tutti e sempre. Il PD, fin dalla scorsa legislatura e anche nell'attuale, sostiene questa esigenza, che va nella direzione vera e garantista del rispetto dei diritti, senza però secondo noi - che questo rispetto confligga con l'interesse generale che hanno tutti i cittadini di rispetto della legalità. Detto questo, l'idea che il pubblico ministero nella sua attività investigativa venga dipinto come una figura oscura fuori controllo, che si impossessa dei dati e non vigila sulla loro divulgazione, per me è malata. Colpire errori, casi colposi o, peggio, dolosi di divulgazione indebita di dati è doveroso; colpire però una categoria intera come la magistratura è tipico di sistemi *(Applausi)* che si possono chiamare in modi diversi, ma certamente non democratici, perché in quelle realtà agli attacchi seguono quasi sempre provvedimenti di sottomissione. A nostro giudizio, questo atteggiamento si configura come una continua opera di delegittimazione della figura del pubblico ministero, che si vuole a tutti i costi rappresentare come estranea alla cultura della giurisdizione, magari con la pericolosa chimera - sì, chimera pericolosa, almeno per me - della separazione delle carriere. Voglio fare doverosamente un riferimento. Anche a me, nel mio piccolo, è capitato, avendo seguito in questi anni i temi della giustizia, di polemizzare con certi atteggiamenti sopra le righe di alcuni pubblici ministeri, con alcuni atteggiamenti iperprotagonisti, con alcuni atteggiamenti che forse potevano sembrare non coerenti con un principio sacro, che è quello del rispetto della presunzione di innocenza. Detto questo, vorrei ricordare che ci sono tanti magistrati e tanti pubblici ministeri che hanno passato la loro vita a combattere i poteri criminali e le mafie, e che per questo vivono sotto scorta. Uno di questi si chiama Roberto Scarpinato e vorrei dire al senatore Renzi che bisognerebbe criticare, polemizzare, ma portare rispetto nei confronti di queste persone per quello che fanno e hanno fatto per tutti noi.

rafforzando ancora di più il ruolo delle difese, senza pregiudicare però la tempestività dell'attività investigativa che - come tutti sanno - ha bisogno di essere svolta con immediatezza, senza intralci burocratici e senza imposizioni anticipate di *discovery* degli atti in fasi ancora delicate, con il rischio di insabbiamento insabbiamento delle prove e di vanificare l'esito di indagini delicate. Sì, il rischio reale è quello di rendere le indagini più difficili, più macchinose. Il meccanismo rischia di diventare un vero e proprio labirinto con due successive autorizzazioni del con i due provvedimenti peraltro impugnabili entrambi al tribunale del riesame e poi in Cassazione. Allungare i tempi prevedendo la doppia procedura di sequestro degli *smartphone* e dei sistemi informatici è una sorta di udienza stralcio che rischia di far disperdere in particolare il materiale archiviato in *cloud*, con un doppio svantaggio: non tutelare affatto i diretti interessati e creare ulteriori difficoltà agli investigatori. Inoltre, si aumenterebbero le difficoltà degli uffici del gip, in quanto si scaricherebbe lì l'onere di controllo sulle acquisizioni dei tabulati. Senza contare poi che aggraverebbe il contesto la previsione di un collegio di giudici - di là da venire peraltro - per decidere le eventuali misure cautelari. Insomma, si è andati molto oltre, ben oltre la sentenza della Corte che chiedeva il rispetto dei criteri di necessità e di proporzione; e ciò anche perché, derogate alcune ipotesi di reato, a cominciare dalle circostanze legate alla criminalità di ordine mafioso e al terrorismo, non si capisce, o forse si capisce fin troppo, il motivo che ha spinto maggioranza e Governo a non considerare, tra le deroghe automatiche, anche quelle riferiti riferite contro la pubblica amministrazione e di corruzione. Signor Presidente, ho concluso. Noi saremmo davvero tentati di votare contro questo provvedimento, non per la sua ispirazione originaria, ma per questo pasticcio. Ma è la prima lettura, questa, e ci aspettiamo che alla Camera le proposte, gli emendamenti, gli argomenti che l'opposizione ha presentato e che qui avete respinto possano invece conoscere un ripensamento. Per questo motivo, non voteremo contro né ovviamente a favore, perché vogliamo ancora credere che su certi temi delicati come questi, che tengono insieme *privacy*, ma anche legalità, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e diritti della difesa, la seconda lettura prossima nell'altro ramo del Parlamento possa essere diversa. Devo essere sincero. Non siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire, ma il PD vuole essere una forza d'opposizione seria, che non vuole rassegnarsi a dire solo no e che fa opposizione indicando alternative a una linea del Governo spesso troppo troppo pasticciata e, in molti casi, dannosa per l'Italia.

da ultimo, alla dichiarazione di voto del Gruppo Fratelli d'Italia su un provvedimento che giudichiamo molto importante per una serie di motivi, che sono già stati in parte anche elencati da chi mi ha preceduto nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto, ma su cui vorrei tornare. Come evidenziato in

sul sequestro degli strumenti informatici, telefonini e *smartphone*, che fanno parte della nostra vita. Questa lacuna ha rilevato come

interpretando quello che è stato scritto, ha evidenziato come, ogni volta che si addiviene al sequestro di un telefonino o di uno *smartphone*, si ha un sequestro smisurato rispetto alla prova che è lo scopo che è lo scopo delle indagini per cui si dispone il sequestro. Oggi la maggioranza è allargata rispetto alle dichiarazioni di voto. Oggi, la maggioranza politica, allargata ad altri settori di questo Parlamento che hanno già annunciato il loro voto favorevole sul provvedimento, ha pensato che fosse necessario intervenire; e lo ha fatto con un'istanza propria, parlamentare, non seguendo *Diktat* o provvedimenti che arrivano dal Governo, come è stato insinuato.

con ricordi indelebili che per alcuni sono solo a loro interno. C'è la vita dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri parenti, di persone estranee alla nostra vita, perché magari nostri clienti o per caso con noi coinvolti. Ci sono le nostre risorse economiche. Ci sono le *password* di tutto quello che serve oggi per vivere. Quindi, è molto di più. Nella discussione si è detto che sequestrare un telefonino è come sequestrare un appartamento. È molto di più, perché in 500 giga di memoria all'interno di un telefonino c'è molto di più, anche di una casa di 500 metri quadrati. Questo perché ci sono beni immateriali che in casa non si trovano, con altre problematiche che oggi noi non abbiamo toccato, ma su cui bisogna riflettere. Quando, infatti, i 500 giga non bastano, noi facciamo riferimento a contenitori esterni di memoria, che non sempre sono situati nel nostro territorio nazionale. E questo è un problema ulteriore, quando si va alla ricerca di notizie dentro i nostri telefonini. Sono soddisfatto e siamo soddisfatti che oggi si arrivi all'approvazione di questo provvedimento che rafforza le garanzie del cittadino, che noi dobbiamo principalmente cittadino che - come è stato detto - è innocente fino al terzo grado di giudizio e così deve essere considerato; cittadino le cui libertà e prerogative non possono neppure essere sacrificate perché questa legge,

siccome forse rallenta e siccome, forse, per dare piena attuazione alla legge ci vorrebbero più magistrati, la libertà di noi cittadini debba rimanere compressa.

di inserire granelli, pietroline, ghiaia o scogli nella macchina giustizia per non farla più funzionare. Non è questo l'intento di chi ha proposto il disegno di legge e non è questo l'intento di chi vota convintamente a favore. L'ho già detto precedentemente: noi siamo uomini liberi, noi siamo donne libere nel nostro complesso. Siamo una maggioranza allargata e libera

Trovo sconcertante che ogni volta che un nostro provvedimento sulla giustizia non piace a qualcuno, venga detto che noi siamo nemici della magistratura. Non può essere, questo rapporto: siccome non fate come diciamo noi, vi ponete immediatamente in contrasto alla magistratura. *(Applausi)*. Non è questo il fine di questa legge. non abbiamo voluto dire e non vogliamo sostenere che i pubblici ministeri non siano in grado di difendere le nostre libertà. Noi vogliamo dire che due persone possono valutare meglio di una. Ma, per garantire comunque le indagini è sempre possibile, laddove le necessità di urgenza lo rilevino, che anche il pubblico ministero possa addivenire al sequestro.

Questo ci riporta a dire che quello al nostro esame non è un provvedimento ideologico, come qualcuno ha voluto sottolineare. Apprezzo anche che il Partito Democratico abbia deciso di astenersi, proprio - io lo interpreto così - perché non ha una posizione ideologica. Probabilmente aveva una posizione differente ma non ideologicamente avversa. Devo dire anche che rifuggo e rifiuto - e rifiutiamo tutti assieme - l'accusa di attuare un garantismo selettivo a favore di qualcheduno.

un'ideologia selettiva nei confronti di qualcheduno o di qualche settore della nostra società o del nostro Stato. I nostri provvedimenti vogliono essere uguali uguali per garantire i princìpi e le libertà di ciascuno di noi, di ciascun cittadino e cittadina italiani.

Ancora una volta mi trovo obbligato a dire che noi rifiutiamo l'etichetta di garantismo classista nei confronti di qualcheduno. Come ho già detto un'altra volta, questo è un linguaggio che si usava negli anni '70 e che fortunatamente è stato superato. Continuare a usare queste queste definizioni, che hanno molto a che fare con la politica e poco con la giustizia, non può essere da noi accettato. Noi, per definizione stessa del nostro movimento politico, rifuggiamo il classismo; non ne parliamo, non lo attuiamo mai e non vogliamo che nessun altro ci metta in bocca di essere classisti, perché così non è. Per noi l'ultimo dei cittadini è il primo dei cittadini e il primo dei colletti bianchi è l'ultimo dei cittadini: per noi non cambia nulla. Noi abbiamo un bene prioritario da difendere, che è quello della buona giustizia e della libertà di ciascuno di noi. E siccome rifiutiamo di essere definiti malintenzionati, con molte buone intenzioni e da benintenzionati votiamo favorevolmente al provvedimento,

riconoscere il ruolo di colui che ha consentito, nel tempo, che la cucina italiana fosse apprezzata in tutto il mondo e fosse considerata oggi, grazie al lavoro svolto nei vari settori che poi elenchiamo nel provvedimento stesso,

di portare, con il grande lavoro che svolgono gli agricoltori, il cibo sulle nostre tavole: un cibo sano, un cibo che si caratterizza per mille provenienze, per caratteristiche peculiari date anche da condizioni pedoclimatiche diverse del nostro Paese, in sostanza

Con questo premio andiamo a riconoscere il grande lavoro del maestro della cucina italiana. Il disegno di legge n. 1010 reca disposizioni per l'istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». L'atto è stato approvato in prima lettura alla Camera, con l'Atto Camera 1419, il 31 gennaio 2024 e trasmesso il successivo 1° febbraio al Senato. Le finalità principali della proposta - di cui all'articolo 1 - sono il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana mediante l'azione del del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità. L'articolo 2 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio «Maestro dell'arte della cucina italiana», conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. L'articolo 3 indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia. L'articolo 4 precisa che il premio è costituito da una medaglia di bronzo. L'articolo 5 stabilisce i requisiti per la candidatura, tra i quali l'aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. L'articolo 6 regola l'*iter* di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno. L'articolo 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 10 stabilisce che l'insignito del premio, il quale si renda indegno, incorre nella revoca dello stesso. L'articolo 11 prevede che, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della proposta in esame, conferisca sei premi di maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3, e che i maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge. è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, identificando la relativa copertura. Ebbene, in conclusione, è evidente che

ma implica aspetti legati alla professionalità, alle capacità, ma anche alla cultura, alla storia, alla tradizione, a quanto il cibo, a quanto l'arte della cucina siano elementi di socializzazione, valorizzazione e apprezzamento del prodotto italiano. Vi è, però, anche un aspetto, come avete potuto notare, legato alla qualità della persona

italiana. Ringrazio il Governo e la Commissione che si è adoperata in tal senso, nonché tutti i colleghi che si sono impegnati per far sì che si arrivasse a questo punto.

Chiedo ai colleghi di lasciare l'Aula se non sono interessati, così il brusio si attenua e noi possiamo andare avanti. Presidente, Sottosegretario, colleghi senatori, la tutela delle eccellenze italiane è un obiettivo che merita sempre un'attenta riflessione da parte di tutti, perché traccia l'identità stessa del nostro Paese. Un obiettivo che è diventato la realtà di un percorso che, da quando il Governo Meloni si è insediato, abbiamo voluto percorrere con caparbietà e l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana che stiamo approvando lo testimonia e ne rafforza l'*iter*. Quando parliamo, infatti, di sovranità alimentare, che non a caso si è voluta fortemente richiamare nella stessa denominazione del Ministero e che il ministro Lollobrigida, con encomiabile testardaggine, non manca mai di sottolineare, parliamo implicitamente di eccellenze della nostra Nazione. Parliamo con orgoglio e convinzione di un lavoro a 360 gradi di promozione di ogni comparto dell'enogastronomia. Per questo rispediamo al mittente qualsiasi volontà di deridere un premio ai nostri artisti culinari, come pure il goffo tentativo delle opposizioni di ridurlo in maniera denigratoria a una semplice medaglia di cartone. Colleghi, dopo le nostre bellezze architettoniche e storiche, la caratteristica per cui il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo è sicuramente la nostra cucina. La cucina italiana è fatta di materie prime pregiate, per la genuinità degli ingredienti, per la loro lavorazione e per la loro tradizione. Questo è indiscutibilmente vero è certificato; basti pensare che siamo i numeri uno al mondo per la biodiversità in ambito agroalimentare. Siamo il Paese europeo con il maggior numero di prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Possiamo vantare di avere ben 326 prodotti tra DOP, IGP e STG; 527 vini certificati con i bollini DOC,

con l'acquolina in bocca, direi. Di fronte a questi numeri noi abbiamo il dovere, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di difendere il buon nome dell'Italia e promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, perché non solo l'Italia è la capitale a livello mondiale della dieta mediterranea e i suoi benefici sono arcinoti e studiati in campo scientifico e accademico, ma anche perché l'arte culinaria contribuisce a costruire la narrazione del nostro Paese all'estero. Come si faccia ad essere contrari a questo provvedimento resta un mistero. Colleghi, il nostro non è il Paese della pizza o del parmigiano, ma è anche il Paese della pizza e del parmigiano, degli spaghetti e del mandolino. Il nostro Paese è e deve continuare ad essere un grande Paese, capace di capace di esportare i propri prodotti e la propria tradizione culinaria nel mondo, capace di valorizzarne la qualità e promuovere la tradizione. È proprio su questi due concetti che il presente disegno di legge si fonda: valorizzare la qualità, conservare le tradizioni e dare supporto alle professionalità, con l'obiettivo di sostenere e promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana, riconoscendo il lavoro e il merito di chi si fa ambasciatore della qualità della nostra cucina nostrana, perché il merito dei successi e dell'italianità nel mondo è anche dovuto a tutti quei professionisti del settore, agli artigiani del cibo, del vino e dell'olio, che ogni giorno nelle loro attività trasformano ed esaltano questi straordinari prodotti e rendono onore al nostro Paese e alla sua fama internazionale. Vogliamo quindi dare un giusto riconoscimento a chi porta avanti la tradizione, a chi tutte le mattine si alza e apre un ristorante, un laboratorio di pasticceria o una gelateria tra mille difficoltà, perché rappresentano l'impalcatura, l'ossatura economica, sociale e culturale del nostro Paese, che ha permesso a tutto il comparto dell'enogastronomia di diventare *leader* mondiale in eccellenze enogastronomiche. Di fronte ad una minoranza che probabilmente preferisce parlare di carne sintetica, di carne coltivata o di farina di grilli, la nostra risposta non può che andare in senso ostinatamente opposto. Noi preferiamo - e lo ribadiamo a gran voce - i prodotti tipici originari, quelli della nostra tradizione, e vogliamo premiare chi lavora a questi prodotti. l'istituzione di questo premio non è altro che una vicinanza delle istituzioni, del Governo e di questa maggioranza, che vanno a stabilire un criterio e a valorizzare ancora di più quella che non solo è una professione, ma una vera e propria arte, perché abbiamo persone che ci mettono cuore, passione e fatica ogni giorno e riescono a portare il *made in Italy* in tutti i Paesi del mondo. Nel merito, con l'istituzione di questo premio vogliamo infatti celebrare il genio italiano dell'arte culinaria, valorizzando la cucina italiana fatta di saperi e di sapori che nulla hanno a che vedere con il cibo spazzatura,

promuovere la nostra cucina significa quindi promuovere il nostro Paese, senza se e senza ma; promuovere la nostra cultura e la nostra identità. Per tutte queste ragioni, annuncio con profondo orgoglio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE-Coraggio Italia.

prendo con estrema serietà l'importanza della nostra cucina e dei nostri prodotti agroalimentari. Ho avuto l'onore di servire la Repubblica come responsabile del nostro commercio internazionale e so bene che gli oltre 50 miliardi che otteniamo dalla vendita dei nostri prodotti agroalimentari sono una colonna della nostra economia e un biglietto da visita della nostra cultura, della nostra impresa, del nostro essere italiani in tutto il mondo. Quindi mi perdoni se il mio intervento sarà severo, perché non vuole in nessun modo sminuire l'importanza della cucina e dell'agricoltura italiana. Signora Presidente, mi lasci dirle una cosa: il fatto che quest'Assemblea sia riunita, peraltro davanti a una scolaresca, per discutere un disegno di legge nell'Aula del Senato dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»" è un segno di grande preoccupazione. Se noi, di mercoledì pomeriggio alle 16,30, non abbiamo da fare nient'altro che questo e - lo segnalo sempre alla povera scolaresca - stiamo per andar via, perché poi non abbiamo più nulla da fare e domani non ci sarà Aula, questa è una dimostrazione preoccupante non per il Parlamento, ma per il Governo che non produce atti legislativi da portare all'attenzione del Parlamento. *(Applausi)*. Perché la verità è che il Parlamento sarebbe ben felice di lavorare, ma la maggioranza, evidentemente, non è in grado di produrre, forse per mancanza di accordi, forse per mancanza di idee, forse per mancanza di politiche, provvedimenti legislativi di una certa serietà. Questo disegno di legge è tra l'altro di iniziativa governativa, non è un disegno di iniziativa parlamentare. Tenete conto, cari ragazzi, che il Consiglio dei ministri si è riunito ha detto: signora Presidente del Consiglio - anzi, signor Presidente del Consiglio - vorrei sottoporre un disegno di legge di iniziativa governativa dal titolo: "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»". Un disegno di legge talmente fondamentale che il costo a carico del bilancio dello Stato è di 2.000 euro. In quest'Aula c'è ora un certo numero di senatori - non so quanti siamo, ma potremmo essere qualcuno di più - che stanno tutti a deliberare su 2.000 euro,

«agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui» si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto (...), «allo scopo parzialmente utilizzando utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste». Immagino si sia riunita anche la Commissione bilancio per dirci, come ha detto il relatore, che l'articolo 12 del disegno di legge individua gli oneri a carico dello Stato e le relative coperture. Complimenti: avete trovato la copertura su 2.000 euro! Peccato che poi qui arrivi un DEF, come leggiamo dai giornali, privo dell'indebitamento programmatico. Non siamo, cioè, in grado di sapere come saranno gestite le finanze pubbliche di questo Paese. Gli investitori non sanno quanto ci dovremo indebitare, ma, grazie al cielo, la maggioranza di destra ha trovato la copertura di 2.000 euro. Io non so veramente come ringraziarvi, perché davvero la solidità delle finanze pubbliche riposa in buone mani.

per assumere trenta nuovi collaboratori. Il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare...

contribuito a scrivere questo pregiato disegno di legge del valore di 2.000 euro. Immagino che ci sia costato di più pagare il collaboratore dell'ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura. Signor Presidente,

Noi abbiamo il tema della peste suina, che è arrivata in un'altra Regione dove prima non era presente e a me piacerebbe poter parlare con il sottosegretario La Pietra di tale questione. Che lui sia bloccato qui

quella che sembra una cosa scherzosa o ironica non lo è. Signor Sottosegretario, questo è un tema politico fondamentale. Perché se questi sono i vostri contenuti, se il vostro Ministero, con tutto quello che c'è dietro (gli uffici e gli esperti) partorisce questo pezzo di carta, io da parlamentare di questo Paese devo essere preoccupatissimo. Ma mi chiedo, che cosa fate lì? Di che cosa vi occupate? Vi occupate di politica agricola comune? Come è possibile? Questo è un sintomo di una crisi decisionale drammatica unita al fatto che, appunto, non producete nelle Commissioni. Se noi oggi non abbiamo più niente da fare e domani non avremo altri disegni di legge da esaminare, vuol dire che l'iniziativa legislativa di questo Governo non esiste, che la proposta politica, la visione del Paese non esiste. *(Applausi)*. La vostra visione del Paese si esaurisce nel premio di maestro dell'arte della cucina italiana. Lo capisce questo? Comprende la gravità politica di questo problema? Non è tanto il disegno di legge, è che cosa questo disegno di legge dimostra: che voi ci teniate in Aula a discutere di questo, dimostra che questo Governo non esiste, non ha un'idea di Paese, non ha un progetto o una visione, oltre a non avere i numeri della finanza pubblica. *(Applausi)*.

e voi ci convocate in Aula, in plenaria, per una legge da 2.000 euro? *(Applausi)*. Signor Sottosegretario, ne tragga le conseguenze politiche.

Senatore Scalfarotto, per la precisione non è vero che domani la Camera e il Senato non lavorano. Domani mattina ci sarà il sindacato senatore De Carlo, so fare il mio lavoro. Domani mattina ci sarà il sindacato ispettivo, domani pomeriggio ci sarà il *question time*, che sono attività primarie delle Camere. Non c'è soltanto l'attività legislativa, ma c'è anche quella conoscitiva e quella di controllo. *(Applausi)*. **Saluto ad una rappresentanza

Quella che a prima vista potrebbe apparire una iniziativa marginale ha in realtà uno scopo importante, cioè quello di ribadire il sostegno delle istituzioni italiane nella promozione delle eccellenze dei nostri territori. Il prodotto italiano rappresenta infatti anche un patrimonio culturale straordinario, che si tramanda e si preserva di generazione in generazione. Parliamo delle nostre tradizioni, dei valori della italianità, realizzati dal lavoro di migliaia di artigiani e imprenditori che costituiscono il meglio della produzione e dello stile di vita italiano. Quindi parliamo di prodotti italiani di qualità, tradizione e sapere, uniti all'innovazione nel modo di produrli, con grande attenzione al momento della socialità. Il loro consumo è di fatto un vero e proprio modello italiano nell'arte culinaria ed enogastronomica e costituisce la dieta mediterranea. Una ricchezza che va

sui mercati mondiali. Vale ricordare che l'Italia possiede il più alto numero di prodotti identificati e garantiti per il tipo di lavorazione e per il territorio dal quale provengono. Il successo di questi manufatti è dovuto alla capacità professionale di tanti esperti, cui è indirizzato il premio che viene istituito con questo disegno di legge. Non solo cucina, ma anche gelateria, pasticceria, arte vitivinicola, olivicola e casearia. Queste sono le categorie in cui ogni anno un maestro per ogni categoria potrà fregiarsi del titolo e dell'apposita medaglia conferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri: un riconoscimento all'unicità e riconoscibilità di alcuni prodotti italiani che sono eccezionali ambasciatori nel mondo. Noi riteniamo che le parole "medaglia di bronzo" vadano intese semplicemente come "medaglia" e che il ministro Lollobrigida vi possa tranquillamente porre rimedio nel primo provvedimento utile. Il premio rappresenta infatti il massimo riconoscimento in quella categoria e va inteso come tale, a prescindere dal materiale con cui verrà coniata la medaglia. Del resto, il provvedimento si inserisce in una serie di disposizioni con cui si è inteso valorizzare e promuovere l'eccellenza italiana, in un percorso normativo coerente. Tra questi ricordiamo il fondo per la sovranità alimentare, istituito con la prima legge di bilancio di questo Governo, dove è presente anche la norma per la promozione del consumo all'estero dei prodotti nazionali di qualità e dove è stato istituito il fondo per la protezione nel mondo per indicazioni geografiche italiane, agricole e alimentari del vino e delle bevande spiritose. Quindi una unità di propositi del Governo Meloni per valorizzare il meglio del meglio dell'Italia creativa e produttiva in campo agroalimentare, cui va il plauso e il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Signora Presidente, rivolgo un saluto alle colleghe e ai colleghi senatori e ai membri del Governo presenti. L'Assemblea, come abbiamo visto in maniera anche abbastanza animata, è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge recante "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»", un provvedimento che - lo dico subito anch'io, Presidente - di fatto non apporta nessuna innovazione e nessuna miglioria sostanziale al mondo della cucina italiana. Un altro, ennesimo, inutile specchietto per le allodole. Guardi, Presidente, noi non siamo contrari a priori a un intervento legislativo in materia, ma sicuramente reputiamo più opportuno un atto amministrativo del Dicastero competente, per ragioni di economia procedurale delle Camere e per una questione di ipertrofia legislativa. Sicuramente troviamo alquanto bizzarro che uno dei settori più importanti dell'economia italiana diventi oggetto di attenzione del Ministero competente solo ed esclusivamente rispetto a interventi pubblicitari, perché di questo alla fine si tratta. Vorrei entrare anche nel merito del provvedimento, nonostante si faccia fatica a trovare questo merito. Provo a fare una sintesi, Presidente. Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio, attribuito da un comitato di selezione nominato da alcuni esponenti dell'Esecutivo, nominati a loro volta tramite decreto del che si rendono noti per le loro qualità culinarie. Ora, Presidente, con tutta la buona volontà e con tutte le buone intenzioni, il Parlamento può veramente esaminare provvedimenti di questo spessore, in un momento storico in cui ci troviamo dinanzi a sfide globali decisamente più importanti e decisamente più urgenti? Avrei compreso e avremmo apprezzato un provvedimento legislativo all'interno del quale, al netto dell'istituzione di questo premio, fosse previsto quantomeno un intervento correttivo delle diverse storture o anche di una sola stortura presente all'interno della filiera della ristorazione. Forse il ministro Lollobrigida e la presidente presidente Meloni non hanno letto l'ultimo *report* sul tema, ma il 2023 è stato un anno nero proprio per la ristorazione. Il numero delle imprese che hanno cessato l'attività, che sono fallite o risultano inattive, ha oltrepassato la vetta delle 28.000 unità e a farne le spese sono le città del turismo per eccellenza, Firenze prima tra tutte, seguita da Roma, Milano, Napoli, Torino. Stiamo assistendo ad una decrescita preoccupante, pericolosa. Le attività di ristorazione stanno diminuendo, con il risultato che più di un ristorante su 100 ha chiuso i battenti. E, se pochissimi anni fa la colpa la si poteva attribuire al Covid, alla significativa diminuzione dei volumi di clientela, adesso non ci sono più scusanti che tengano. La situazione non è migliore neanche sul versante dei bar, un'altra espressione di italianità nel mondo, con i suoi prodotti di pasticceria e e bevande iconiche: pensiamo al cappuccino, al caffè espresso. Dopo cinque anni solo un bar su due riesce a restare sul mercato. I dati del primo semestre del 2023, poi, mostrano come anche in questo caso le chiusure oltrepassano in maniera significativa le aperture di nuove iniziative imprenditoriali. Su poco più di 1.100 piccole aziende che fanno capolino, infatti, ve ne sono più di 1.008 che chiudono per sempre le porte di entrata. Ecco perché occorre un immediato piano d'azione supportato economicamente per sollevare un settore che sta precipitando, non certo delle medaglie, tra l'altro pure di bronzo. Confortante sarebbe stato assistere ad una politica di coordinamento tra le imprese della ristorazione e gli istituti alberghieri, ad esempio favorendo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro su meccanismi lavorativi; oppure ragionare su un provvedimento legislativo che intervenisse sulla carenza di personale, sulla previsione di strumenti anche di agevolazione fiscale, che incentivasse assunzioni, stabilizzazioni del personale o ancora l'istituzione di istituti tecnici superiori che favorissero la creazione e la strutturazione di figure professionali necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni - quelli veri - del settore della ristorazione. Utile sarebbe stato prevedere strumenti di agevolazione delle imprese impegnate nel settore rispetto all'assunzione di giovani, incidendo sul lavoro povero, sulla precarietà, sulla difficoltà dei lavoratori stagionali, perché vi do una notizia: quello che questa maggioranza interpreta come aumento dell'occupazione

puntando ad un mercato del lavoro più precario e con sempre meno tutele. Non c'è stato un intervento legislativo che sia uno di questo Governo volto a superare le difficoltà della nostra economia. Ma come si fa ad essere soddisfatti, ad essere orgogliosi davanti alla crescita pari a zero, davanti all'aumento delle disuguaglianze? Ma che dati leggete? La politica di questo Governo non risolve, addirittura aggraverà i problemi, perché non può essere diversamente se si comprimono i salari, se si aumenta la precarietà. Sapete quale lavoro sta aumentando e per il quale avete esultato? Quello sottopagato, quello che per forza, per disperazione bisogna accettare, accettando così di diventare lavoratore povero. Però ci sono le medagliette, e va bene. Questo segmento dell'economia mai come ora avrebbe avuto bisogno di una sana boccata di ossigeno, perché troppi sono stati gli imprevisti duri vissuti da questo settore: una pandemia mondiale, la crisi del personale, l'inflazione e i rincari energetici. Politiche pubbliche non dico perfette, ma sensate, utili: è di questo che c'è più che mai bisogno, non di sorrisini, pacche sulla spalla, medaglietta istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inutile e non funzionale alla risoluzione delle problematiche inerenti il settore della ristorazione. Ma lo sappiamo: voi siete continuamente in campagna elettorale e, quindi, via libera a questi provvedimenti in pieno stile *spot* pubblicitario. Se c'è una filiera che nel nostro Paese, con questo Governo, non conosce crisi, Presidente, è quella della fantasia legislativa marginale e superflua. Oggi potremmo consegnare addirittura una medaglietta d'oro. Per tutte queste ragioni, coerentemente con la posizione assunta dai colleghi del MoVimento 5 Stelle alla Camera, annuncio il voto contrario a questo provvedimento. Signor Presidente, oggi è in approvazione un disegno di legge per l'istituzione del premio al merito di Maestro dell'arte della cucina italiana, rivolto ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia, nelle categorie della gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura, arte casearia, e con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana facendo conoscere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana nel mondo. Come correttamente recita il provvedimento, l'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività e questo è un passaggio fondamentale.

provvedimento che ha istituito un premio volto al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità. Il premio annuale - è vero - è costituito da una medaglia di bronzo con l'emblema della Repubblica italiana e la dicitura relativa alla categoria,

Io con molti colleghi che vedo qui mi sento responsabile della mia azione in Commissione e in Aula, perché ci sono e credo che questo sia importante; senatrici e senatori meritano moltissimo rispetto, perché lavoriamo perché lavoriamo tantissimo. Perciò, signora Presidente, certi atteggiamenti non sono solo deplorevoli, ma vanno a inficiare il prezioso lavoro di molte persone qui in Senato. - come stavo dicendo - si inserisce in un quadro normativo volto a sostenere, promuovere e tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, che ha già visto l'incremento di 200.000 euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, volto a promuovere e sostenere

istituito il Fondo per la sovranità alimentare, volto a rafforzare il sistema agricolo nazionale, con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026. Infine, la legge di bilancio 2024 ha disposto il rifinanziamento di alcune misure volte al sostegno degli indigenti, per gli acquisti di beni di prima necessità, stabilendo l'incremento di 600 milioni di euro solo per quest'anno del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburante e di abbonamenti istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sulla tutela del *made in Italy*, ricordo a tutti i colleghi che questo disegno di legge in quel provvedimento, la legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, che include la certificazione della ristorazione italiana nel mondo, sulle misure di promozione della cucina italiana all'estero, nonché sull'istituzione di un fondo per la tutela delle indicazioni geografiche registrate dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo.

ed anche il fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche protette. Sappiamo che l'*italian sounding* è uno dei problemi enormi che ha il nostro prezioso prodotto italiano, il nostro *made in Italy* che con tanta fatica viene prodotto dai nostri agricoltori, dai nostri produttori agricoli. Credo che l'impegno il sostegno dell'agroalimentare italiano per la tutela della salute passi anche attraverso il conferimento di premi a coloro che svolgono questo lavoro con fatica e valorizzano un settore così fondamentale della nostra economia. Negli ultimi anni siamo stati attaccati da parte del resto del mondo, in particolare da parte dell'Unione europea. C'è stato un attacco feroce alla dieta mediterranea e questa è anche una risposta; così come abbiamo risposto approvando una legge che dice che l'agricoltore è custode dell'ambiente e del territorio. Allora, anche qui, la capacità di definire e istituire il premio di maestro di arte della cucina italiana valorizza un'altra parte importante della filiera dell'agroalimentare italiano. È di questi giorni, Presidente, la protesta di Coldiretti, che è partita con una mobilitazione al valico del Brennero per una proposta di legge europea sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola: chiede l'obbligo di etichettatura di origine dei prodotti europei, ma anche di abolire la normativa relativa alla lavorazione sostanziale garantita dal codice doganale, per contrastare il proliferare del fenomeno dell'*italian sounding*, che spaccia come italiani prodotti lontani dalla nostra storia e dalle nostre tradizioni, nonché di qualità scarsissima. Noi vogliamo il principio di reciprocità: chi porta anche solo 10 grammi di prodotto alimentare in Italia, questo deve essere prodotto con le stesse caratteristiche con cui gli italiani lo producono. *(Applausi)*. Non possiamo più permetterci che non ci sia un principio di reciprocità questo lavoro lo stiamo facendo in Commissione e lo faremo anche la prossima settimana, quando daremo il parere sulla Politica agricola comune. È indispensabile incrementare anche i controlli per bloccare le truffe a tavola. Dobbiamo dire basta all'importazione di prodotti che usano sostanze vietate che poi ci vengono propinate. Ma gli attacchi inferti dall'Europa non si fermano: a dicembre c'è stato l'attacco della Corte dei conti dell'Unione europea nell'*audit* sui decreti italiani sull'etichettatura d'origine;

Ricordo che almeno otto italiani su dieci chiedono lo stop alle importazioni di prodotti alimentari che non rispettano le stesse regole di quelli italiani. Assurdo poi che l'Unione europea si rifiuti di fare chiarezza su prodotti che incidono fortemente sull'economia di una Nazione, *in primis* sulla salute dei suoi cittadini. Anche qui ricordo che la nuova PAC punta sulla sostenibilità, ma a spese degli agricoltori, che in realtà sono i primi ambientalisti del pianeta. Per questo, signora Presidente, è importante continuare a combattere per difendere la qualità delle nostre produzioni, la trasformazione in tavola, il lavoro delle nostre aziende già piegate dalla crisi climatica ed economica, dalle pesanti ripercussioni delle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. i riconoscimenti rivolti a coloro che sono custodi e ambasciatori di questo valore inestimabile e delle eccellenze culinarie italiane cadono nel momento giusto e trovano riferimento nel lavoro compiuto con dedizione e passione dai nostri cuochi, che anche qui definirei i custodi dell'eccellenza agroalimentare italiani. *(Applausi)*. Signora Presidente, lo diceva Tolstoj: solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale e morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario, essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra sempre:

che la cucina non sia un'arte, una storia, una cultura, una tradizione, un valore turistico, culturale e identitario delle nostre tante Regioni e del nostro Paese nella sua interezza.

perché qui di collegamenti con la filiera, con la salvaguardia della sostenibilità produttiva, del chilometro zero e dell'identità territoriale non c'è nulla.

aver maturato quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza; aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. Dove sono tutte le misure di sostegno all'agricoltura che sono state narrate fin qui? Questo provvedimento, infatti, ben si collocava rispetto a quello che è stato detto, cioè la valorizzazione della filiera. Sappiamo tutti che oggi uno dei più grossi problemi che ha l'agricoltura italiana è la differenza tra quello che viene pagato all'agricoltore e il costo del prodotto sullo scaffale o al ristorante. *(Applausi)*. Allora bisognava valorizzare la filiera anche ai fini dell'ottenimento di un riconoscimento che avrebbe avuto una specificità e una particolarità. Si parla di Si parla di settore, come ho sentito anche in altri interventi. Oggi la ristorazione ha tanti problemi. Uno dei principali problemi è la formazione professionale, ma troppo spesso nei nostri provvedimenti non vediamo inserite quelle condizioni di formazione professionale di base, che siano gli istituti professionali, nella fattispecie l'alberghiero, o le agenzie formative che dovrebbero fare gli istituti professionali per formare personale che poi deve andare a lavorare in quei settori che hanno una forte caratterizzazione, una forte specialità. Anche questo nel provvedimento non lo troviamo. Si tratta di un disegno di legge che purtroppo

Noi non ci sentiamo di votare uno *slogan*; noi vogliamo votare dei contenuti. Se si voleva dare un premio, oltre a sostenere giustamente il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia alimentare e dell'agroalimentare, istituito nel 2022 dal Governo Draghi, e non con 200.000 euro euro ma con molte più risorse che sarebbero necessitate per questo tipo di sostegno, oggi, per contro, ci troviamo solamente a definire un premio che è una medaglia di bronzo

noi riteniamo di dover impiegare il nostro tempo in altro modo. Noi siamo ben fieri di stare qui e di servire il Paese con gli atti che si necessitano, ma gli atti sono di varia forma e di vario contenuto

è legislativo. Se questo premio aveva raggiunto l'obiettivo per il quale era stato posto, potevano essere apportati i giusti correttivi in modo molto più snello e molto meno burocratico senza impegnare i due rami del Parlamento per un disegno di legge che, una volta fatto, assume un valore completamente diverso da un atto amministrativo. *(Applausi)*. Questa è una contraddizione anche rispetto a quanto diciamo e sentiamo nelle campagne elettorali. Anche quando abbiamo affrontato il tema dell'agricoltura alla presenza della Presidente del Consiglio dei ministri, uno dei punti era la burocrazia. Ma come si fa a chiedere la sburocratizzazione del Paese quando noi siamo i primi burocrati che costruiscono norme che si potevano fare in altro modo,

noi siamo fieri di tutte le maestranze, dei cuochi e di tutti coloro che lavorano nelle cucine, che tengono alto l'onore in Italia e all'estero, perché la cucina italiana è un valore non solo all'interno dei confini nazionali, ma nel mondo. Ma non ce la sentiamo di dar loro un riconoscimento nella forma che viene proposta con questo disegno di legge, perché non è dignitoso dignitoso per la professione che rappresentano. Per questo annunciamo il voto contrario del Partito Democratico.

siamo qui oggi per discutere e approvare il disegno di legge per l'istituzione del premio di Maestro dell'arte della cucina italiana, è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ci stiamo impegnando costantemente e instancabilmente per mettere ogni giorno la promozione del nostro patrimonio enogastronomico

valorizzare e difendere un patrimonio unico e inimitabile, qual è la nostra cucina italiana. fino al punto da avanzare la proposta di riconoscere la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità, dell'UNESCO. Sappiamo tutti quanto la cucina italiana rappresenti un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, come sono conosciuti i prodotti *made in Italy* di altissima qualità e le ricette storiche che per ogni Regione d'Italia hanno la propria identità e tradizione.

dei cuochi italiani, che rendono la nostra cucina italiana famosa e invidiata a livello internazionale. Con questo provvedimento si è voluto creare un riconoscimento per i grandi talenti italiani che fosse tutto italiano, un premio per i maestri di cucina e di pasticceria. Il simbolo di questo premio è proprio il maestro pasticciere Igino Massari. Della nostra cucina dobbiamo essere orgogliosi, ma la cucina nasce anche dalla ricerca delle materie prime che in Italia sono così variegate e di qualità, dalla stratificazione di tante culture e contaminazioni, dalla rappresentazione attraverso alcuni personaggi che si fregiano di una titolarità che gli viene data dalle loro capacità e dalla loro esperienza. Ritengo quindi giusto che un buon Governo debba individuare le persone che nel mondo possano fregiarsi della loro capacità, al pari dei maestri di altre Nazioni, ad esempio la Francia,

quello che la nostra produzione enologica sa valorizzare, quello che la nostra produzione olivicola sa rendere eccellente.

per trasmettere ai giovani la grande tradizione italiana, che spesso deriva dall'esperienza che hanno accumulato e conquistato nel tempo e che è giusto che uno Stato metta a disposizione delle nuove generazioni. Spesso la nostra Nazione difetta della valorizzazione delle professioni tecniche. L'ascensore sociale spesso è legato alla formazione umanistica e la scelta di altre attività è stata considerata di secondo piano. piano. Vediamo che ha effetti anche sull'occupazione, perché tanti ragazzi che hanno scelto il percorso universitario fanno poi fatica a posizionarsi nel mondo del lavoro, quando avrebbero potuto seguire una passione come la cucina e imparare un mestiere. Si tratta molto spesso anche di talenti da coltivare attraverso la cultura, nel mondo dell'arte, dell'artigianalità e, insomma, della creatività. Il Governo Meloni cerca di riavvicinare molto le giovani generazioni ad alcuni maestri che hanno fatto la storia di questa Nazione, che sono l'orgoglio italiano, ma che sono stati disincentivati e che potrebbero ridare grande valore nel futuro al *made in Italy* e migliorare anche di molto i dati occupazionali. Questo va di pari passo con iniziative del Governo in tale direzione, come l'istituzione del liceo del *made in Italy*, come stimolo ad avvicinarsi a queste professioni e a formare e far crescere e far crescere sempre più ambasciatori delle bellezze e delle eccellenze del nostro patrimonio nazionale, come quelli che con questo premio si vogliono premiare e ringraziare. L'auspicio espresso dal Governo e che condividiamo noi oggi in quest'Aula è che anche questa legge possa essere un contributo per omogeneizzarsi in senso positivo ad altre Nazioni dell'Unione dell'Unione europea, che sono partite prima e hanno già raggiunto risultati che noi auspichiamo di contribuire a raggiungere, se non di superare.

Penso valga la pena investire 2.000 euro con trasparenza per questo premio, per raccogliere moltissimo in termini di valore economico e culturale grazie ai tanti talenti che nel tempo hanno saputo valorizzare la nostra Nazione attraverso le loro grandi capacità creative e di ricerca, rendendolo un esempio che oggi, grazie al Parlamento, sarà un riconoscimento istituzionale da parte del Governo. Ricordo infine che sono stati investiti 8 miliardi di euro nei diciotto mesi di questo Governo: si tratta del più grande stanziamento mai fatto prima dai Governi precedenti.

ha fatto personale quando a un senatore vengono attribuite opinioni contrarie a quelle espresse. Il tema era proprio questo ed è quello che ho cercato di fare prima. prima. Io ho fatto un intervento politico e lei, Presidente, ha ritenuto di chiosare il mio intervento, mettendomi in bocca parole che io non avevo detto. Ai fini del verbale, io non ho detto che il Parlamento non lavora; ho detto che il Governo non è in condizione di mandarci disegni di legge da approvare

con grande franchezza e grande tranquillità, che non mi sono sentito garantito, come parlamentare, nelle mie prerogative, che sono quelle di esprimere la mia opinione e di non sentirmi commentare dalla Presidenza, perché la Presidenza dovrebbe avere la caratteristica di essere *super partes*. Lei ha chiosato il mio intervento, volendo l'ultima parola sulle cose che io dicevo. Questo secondo me non è corretto o, quantomeno, mi ha fatto sentire leso nelle mie prerogative, che sono quelle di rappresentare i miei elettori. Se lei toglie la parola a me, la toglie ai miei elettori; io sono qui per rappresentare loro e e rispondere soltanto a loro. Dico un'ultimissima cosa. Vorrei scusarmi molto profusamente nei confronti degli Uffici: se per qualche ragione gli Uffici si sono sentiti tirati per la giacca da me, me ne scuso moltissimo, perché la stima

trova un salvagente dove lo trova. Per questo mi scuso, non accadrà mai più. La Presidenza di turno mi aiuterà a non far accadere questo, se svolgerà il suo compito con quelle caratteristiche di terzietà signora Presidente, lei oggi francamente non ha avuto. secondo l'articolo 90 del Regolamento. Io non ho commentato il suo intervento e vorrei che rimanesse a verbale anche questo. Ho fatto una precisazione. Lei ha parlato di Aula che non lavora e io, in quanto Presidente in questo momento, difendo l'Aula del Senato, che domani lavora. Presidente, grazie. Ho ascoltato, essendo presente in Aula in quel momento, e ritengo che il suo intervento e quindi il comportamento della Presidenza sia stato ineccepibile. Eravamo di dichiarazione di voto ed era già aperto il microfono del collega che stava intervenendo. Lei ha fatto solo un richiamo all'ordine, perché si stava andando oltre. oltre. Non c'è stata alcuna chiosa sulle opinioni politiche che ha espresso liberamente il collega qui in Aula. Io ritengo che il fatto non sussista e che ci sia stato un comportamento corretto da parte della Presidenza.

Signor Presidente, ho chiesto la parola per una cosa che sentiamo molto, ma che credo possa essere nel sentire comune di tutta l'Assemblea. Noi vorremmo abbracciare da qui le famiglie, le fidanzate, gli amici di due ragazzi

sono morti per strada l'altro giorno vicino a Eboli. Stavano lì, il maresciallo Pastore e l'appuntato scelto Ferraro, a difendere la sicurezza di tutti i cittadini. Vorremmo abbracciare anche le comunità di Manfredonia e Montesanto Salentino che ieri hanno dato l'ultimo straziante saluto ai loro figli. Siamo vicini, naturalmente, all'Arma dei carabinieri colpita dalla perdita sul campo di questi due ragazzi che avevano scelto questa strada perché volevano stare dalla parte della legalità. Avrebbero potuto perdere la vita magari perché colpiti da rapinatori, mafiosi, terroristi e sono morti probabilmente lo diranno le inchieste e i giudizi della magistratura - per omicidio stradale. Questo non rende ovviamente meno crudele e doloroso il loro sacrificio, anzi, ma una cosa è certa: ricordiamo tutti che questi ragazzi stavano lì per tutti noi, come fanno ogni giorno tantissimi altri ragazzi in divisa e per questo non li dimenticheremo.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

La seduta è tolta